capisco le critiche di natura economica; capisco meno che si parli di decadenza morale dell'Italia, come hanno fatto oggi i senatori Asciutti e Bonfrisco proprio il giorno dopo il voto dell'ONU sulla pena di morte, dimenticando così che quello di ieri è stato un successo di tutto il Paese, non certo solo di questo Governo. Sono lieto di aggiungere alcune considerazioni favorevoli alla manovra finanziaria per il 2008. Si è parlato, in Aula e in Commissione, come sempre avviene, più della legge finanziaria che della legge di bilancio. Eppure, anche se nella finanziaria si gioca la sorte di più del 97 per cento delle risorse dello Stato, è nella legge di bilancio che quest'anno vi sono state le maggiori novità formali. Il relatore Albonetti ci ha spiegato bene, pur non lesinando alcune critiche, con le parole e con utili tabelle - che valgono assai più delle parole - cosa c'è di nuovo nel bilancio dello Stato: la struttura per missione e, soprattutto, a cosa serve questa novità. Serve, in estrema sintesi, a far capire meglio dove vanno i soldi dei cittadini. Per usare una vecchia parola, serve alla democrazia senza aggettivi. Proprio l'aggettivo mi aiuta ad introdurre il discorso sulla finanziaria in generale ed in relazione alle modifiche della Camera. A scuola ci insegnavano che vi erano i gradi degli aggettivi: i comparativi e due tipi di superlativi. Vi faccio alcune domande utilizzando queste categorie: ci troviamo di fronte ad una legge finanziaria buona? Probabilmente sì. Migliore di quella dello scorso anno? Certamente sì. Quella uscita dalla Camera è migliore di quella uscita da quest'Aula? Quasi sempre sì. È la migliore tra quelle possibili, in relazione alla situazione politica data? Probabilmente sì. È una legge finanziaria ottima, si può usare il superlativo assoluto? Forse no. Per spiegare perché ho parlato di migliore legge possibile oserei paragonare la legge finanziaria ad una torta, fatta di una parte sostanziale e poi ornata di ciliegine e quant'altro. Bene, a mio avviso, il nucleo della torta è stato fatto bene dal Governo e non è cambiato nella sostanza e nei saldi, salvo piccoli miglioramenti nei due passaggi parlamentari. La minoranza ha ironizzato su alcune piccole spese, alcune discutibili nel merito, altre nell'ammissibilità, ma erano ciliegine, magari indigeste, ma quantitativamente, anche sommate tra loro, non rilevanti. Sviluppo alcuni punti. Rispetto all'anno scorso la legge finanziaria è un po' più snella. Si sa che è partita assai più magra ed è uscita di qui un po' ingrassata, ma ancora in buona forma, cioè leggibile, con tutti i suoi circa 150 articoli con la loro rubrica, divisi in Capi corrispondenti a missioni. Dalla Camera è tornata accresciuta e disarticolata ed è tornata ad essere, come negli ultimi anni, una struttura informe, quasi uniformata alle ultime analisi del CENSIS, ma è rimasta più leggibile di quella dello scorso anno. Venendo ai contenuti, rispetto al 2007 la legge finanziaria 2008 si è potuta dedicare di più alla redistribuzione parziale del reddito ed allo sgravio fiscale, dovendo meno dedicarsi al risanamento. Non ci sono nuove tasse, né aumenti di aliquote, tranne minime eccezioni. Questo diciamolo forte, perché sono smentiti i vaticini dell'opposizione. La principale critica dell'opposizione è che il Governo, di fronte a prospettive congiunturali peggiori di quanto si era prospettato nel DPEF, non metterebbe da parte risorse. Tuttavia, anche gli ultimi dati sulle entrate fanno pensare che le prospettive dell'anno prossimo prevedano dei conti a posto. Bisogna infatti considerare, come è stato osservato, anche se non è elegante dirlo, che un limitato aumento di inflazione potrebbe favorire le entrate 2008. La riduzione dell'ICI, l'intervento in favore delle locazioni, il "forfettone" hanno attraversato, con pochissime modifiche, tutto *l'iter* parlamentare. L'anno scorso il succedersi delle soluzioni fiscali aveva creato un percorso di guerra mediatico, che aveva nociuto al Governo più delle soluzioni in sé. La riduzione dell'IRES, assai criticata dall'opposizione (dimentica che questo era uno dei propositi dei primi documenti fiscali del disegno della destra: riduzione delle aliquote e aumento della base contributiva), costituisce probabilmente la principale misura per lo sviluppo, almeno a medio termine. Ne può derivare, sia pure in pochi settori caratterizzati da concorrenza perfetta o quasi, anche una riduzione dei prezzi e credo che forse questa potrà essere per certi aspetti ed in certi settori una misura più efficace di "Mister In questo campo (riduzione dell'IRES), la Camera è intervenuta estendendo l'allineamento della disciplina fiscale a quella del bilancio civilistico anche alle società che adottano i princìpi contabili internazionali. Vorrei aggiungere alcune osservazioni sulla pressione fiscale. È vero che la pressione fiscale, a partire dal 2005, è cresciuta di due punti. L'incremento del 2007 si attesterà su livelli molto simili a quelli del 2006 e comunemente non si considerano due circostanze. In primo luogo, che all'interno della pressione fiscale 2007, tecnicamente in maniera giusta, si comprende anche il trasferimento del TFR al l'INPS, che è sì un trasferimento di denaro dal privato al pubblico, ma non corrisponde ad una diminuzione patrimoniale per chi fa questo versamento. Inoltre, la riduzione del cuneo fiscale incide soltanto su sei mesi del 2007. È altresì necessario osservare che i risultati del 2007 non dipendono da nuove tasse o da modifiche di aliquote, di aliquote, ma sono dovuti ad un recupero di base impositiva, a un recupero di evasione, ad un complesso di attività amministrative e anche alla riforma dell'esazione. poi un curioso atteggiamento nell'opposizione. Probabilmente i buoni risultati del 2007 sono

1, che rende più stringente e vincolante la destinazione dell'extragettito allo sgravio dei redditi da lavoro.

Il primo problema riguarda cosa succede se non si raggiunge il 20 per cento previsto nella norma stessa. Qualcuno ha sostenuto che in tal caso la norma diventa applicabile;

rende certamente più chiara l'applicazione, ma forse può cambiare la platea degli utenti. Ringrazio, dunque,

Le spese sono sotto controllo, il loro incremento è assolutamente limitato e rimane nell'ambito dei parametri previsti dai documenti preparatori della legge finanziaria. Si è anche dato per scontato che vi sia una equivalenza tra aumento delle spese e assunzioni nella pubblica amministrazione.

sembra necessario affrontare il problema dei precari della pubblica amministrazione, uno dei grossi temi su cui è intervenuta la nostra Assemblea. Faccio subito una premessa: nelle polemiche di oggi si è partiti da un presupposto dato per ovvio, che non è affatto vero, cioè che ogni, qualsiasi eventuale assunzione di precari sia supplementare rispetto agli organici della pubblica amministrazione e che

Innanzi tutto, si è stabilito il principio - che avrà poche eccezioni - che, di qui in avanti, non si assumerà più in maniera precaria o, comunque, a tempo non indeterminato. Quindi, si è cercato di fissare un quantitativo di persone e

temo - ritroveremo ad ogni finanziaria. Comunque, si è stabilito un diritto a rimanere dove si è: si è indicato un percorso, rigorosamente basato, però, su formule selettive concorsuali, per un inserimento negli organici della pubblica amministrazione. Prima dicevo che questa finanziaria è buona, la migliore possibile, ma forse non è ottima: si possono fare alcune critiche a questa soluzione? Sì;

un'occasione per favorire, in questa fase del pubblico impiego, una mobilità interna: forse è un'occasione che è stato un peccato perdere. L'ultima osservazione che vorrei fare riguarda una norma, di cui qualcuno ha parlato oggi,

sulla limitazione del Fondo unico

indipendentemente dal conseguimento di effettivi risparmi. La soluzione della Camera interviene su questo punto, prevedendo una verifica sull'effettività dei tagli e quindi una possibile riduzione - scusate

i relatori sul disegno di legge di bilancio e sulla finanziaria hanno dato conto a quest'Aula delle modifiche intervenute in sede di discussione alla Camera

vuol essere un atto di solidarietà nei confronti del ministro Padoa-Schioppa, del vice ministro Visco e del ministro Bersani, fatti oggetto di una minaccia

che quest'Aula, a prescindere da come si giudichi l'operato politico di ciascuno di questi soggetti, esprima la propria condanna nei confronti di questo gesto e la propria solidarietà nei confronti delle persone. La seconda considerazione è in relazione alla denuncia che avevo fatto questa mattina, sulla quale mi auguro che i rappresentanti del Governo siano in condizione di impegnare anche i loro colleghi che hanno una responsabilità diretta

quantomeno fino a quando le strutture dello Stato, della pubblica amministrazione e del Comune di Roma non siano in grado di dare ospitalità e accoglienza a bambini e donne, anche in stato di gravidanza. Fintanto che la nostra pubblica amministrazione, la nostra Repubblica non è in grado di garantire questi diritti elementari non può sentirsi abilitata ad esercitare un potere di sgombero. C'è un problema di civiltà, signor Sottosegretario. La invito a chiamare i suoi colleghi e invito il Presidente a farsene carico. Non è infatti in discussione

redistribuzione delle quote di reddito aggiuntivo prodotte dalla lotta all'evasione fiscale e dall'accresciuta fidelizzazione dei cittadini rispetto al sistema fiscale, che hanno dato luogo a quelli che abbiamo definito, in linguaggio giornalistico, "tesoretti". L'avere avviato una timida redistribuzione significa che ci siamo messi sulla buona strada. Insufficiente, perché questa strada si scontra con una soluzione assolutamente

prestazioni straordinarie detassate, quindi incentivate dal fisco, finiscono bruciati o precipitati

Pretendiamo non soltanto un di più fatto di norme, di capacità di intervento, di aumento delle capacità di intervenire da parte degli ispettorati del lavoro, delle ASL, ma anche il riconoscimento dei poteri di controllo dei lavoratori sulla propria condizione. Infatti, signor Sottosegretario, il problema che spesso viene evocato è quello dei controlli, dell'aumento dei controlli da parte delle ASL e degli ispettorati del lavoro, cosa assolutamente fondamentale,

funzioni di controllo sull'organizzazione del lavoro, sui carichi di lavoro, sulla nocività ambientale, sulle condizioni negative che determinavano la pericolosità di quel posto di lavoro, allora, quando i sindacati dei lavoratori potevano esercitare liberamente e in maniera garantita dallo Statuto dei diritti dei lavoratori quelle prerogative che non sono degli abusi, si è assistito al calo degli incidenti sul lavoro. Da quando, invece, anche il diritto sindacale, l'esercizio dei poteri di rappresentanza sindacale è conculcato in nome della libertà di impresa e della libertà del mercato, non potendo più esercitare questi poteri di autogoverno della forza lavoro, vi è un'esposizione assolutamente esasperata, con una crescita esponenziale degli incidenti sul lavoro, delle malattie professionali e delle condizioni di insicurezza. Dobbiamo rompere questa catena di ricatto, la quale è attivata dal fatto che i salari non coprono i fabbisogni essenziali delle famiglie, vi è ancora una quota consistente di famiglie che non arrivano al limite di sussistenza, un'ampia fascia di persone che non riescono ad arrivare alla fine del mese, mentre quelle fasce di cosiddetto ceto medio si impoveriscono progressivamente. Da questo punto di vista, è importante che nella finanziaria sia stato anche definito il fondo attraverso cui, a partire dal 2008, ci sarà un intervento di alleggerimento del prelievo fiscale sulle fasce basse del lavoro dipendente, a partire dall'abbattimento dall'abbattimento del *fiscal drag*; penso che dobbiamo lavorare e che il Governo debba favorire lo sviluppo della contrattazione sindacale, anche con la definizione del contratto dei lavoratori metalmeccanici, mettendo sul tavolo la defiscalizzazione degli aumenti salariali, perché questi consentono alle imprese e ai sindacati di trovare l'intesa sul rinnovo contrattuale dei lavoratori metalmeccanici.

quello che capisco meno è che da parte del Governo vengano proposti in una Camera provvedimenti che nell'altra non sono stati proposti o, se proposti, sono stati respinti o concordemente accantonati. Da questo punto di vista, trovo che due sono elementi assolutamente inaccettabili; abbiamo risolto, attraverso una mediazione intelligente di cui devo dare atto ai sottosegretari Sartor e Grandi, la questione degli idonei dell'Agenzia delle entrate, per quanto riguarda l'ambiente e i CIP 6 e per quanto concerne l'introduzione nella legge finanziaria del concetto di perequazione urbanistica, trovo che sia una forzatura inaccettabile che il Governo deve impegnarsi a rimuovere, perché non è quella della finanziaria la sede in cui si può intervenire per una nuova legislazione urbanistica nel nostro Paese. Far passare di soppiatto una norma che serve soltanto ad alcuni sindaci spregiudicati e ad alcuni costruttori altrettanto spregiudicati è inaccettabile! *(Applausi dal Gruppo RC-SE).* PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ciccanti. Ne ha facoltà. *(UDC)*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il 13 dicembre scorso il ministro Tommaso Padoa-Schioppa, nel presentare il Rapporto intermedio sulla revisione della spesa pubblica, ha dichiarato: «C'è ancora molta strada da fare nei prossimi tre anni per arrivare al pareggio di bilancio. Servono almeno 30 miliardi di euro nel prossimo triennio per sistemare i conti pubblici. Gran parte della correzione deve avvenire sul lato della spesa, se si vuole che la pressione fiscale non aumenti ancora». Purtroppo, la prima sia questa seconda finanziaria hanno smentito le buone intenzioni professate: la spesa pubblica è cresciuta e la pressione fiscale pure. Per la seconda volta, avete fatto un DPEF che diceva una cosa e una finanziaria che ne dice un'altra. Ancora una volta, il Governo approva un testo del disegno di legge e la maggioranza lo riscrive totalmente. Non riteniamo la centralità del Parlamento una scelta occasionale o un valore costituzionale a geometria variabile, il Parlamento smentisce se stesso, attraverso una maggioranza mutevole negli interessi e negli umori. In questo caso, quando la maggioranza di centro-sinistra, a fine settembre, rivede tutti gli obiettivi di finanza pubblica con la Nota di aggiornamento e la relativa risoluzione e, qualche settimana dopo, la stessa maggioranza li scavalca per esigenze di clientele elettorali, si pone una questione democratica seria relativamente alla credibilità e affidabilità del Parlamento e alla sua centralità rispetto alle esigenze mutevoli del Governo. In tale circostanza, si ferisce la dignità del Parlamento, oltre che la coerenza dei conti pubblici. Voi, colleghi del centro-sinistra, avete sulla vostra coscienza politica questa doppia colpa, che alimenta l'antipolitica e indebolisce la democrazia in Italia. Ma veniamo ai conti della finanziaria e del bilancio. Innanzitutto, per il 2009 e 2010 aumentano le entrate. Il testo approvato dalla Camera, rispetto a quello del Senato, aumenta nel triennio 2008-2010 le entrate di 230 milioni di euro. Rispetto al testo del Governo, emerge un aumento delle entrate di 284 milioni, 378 milioni e 942 milioni di euro, rispettivamente per gli anni 2008, 2009 e 2010. Questo significa anche un aumento della pressione fiscale, per l'aggiunta di quella che si renderà necessaria per raggiungere il pareggio di bilancio, così come il Governo si è impegnato a fare nel 2010 con i Paesi dell'area euro. Per il 2007 la pressione fiscale ha raggiunto il 43 per cento e tale si presume rimarrà nel 2008 a legislazione vigente, anzi, per alcuni osservatori dovrebbe addirittura aumentare. A pagare le tasse sono sempre gli stessi! L'aumento delle entrate che ho citato è il risultato netto tra maggiori e minori entrate, determinate da diverse misure della finanziaria. Quello che è grave è che, secondo lo studio del Servizio bilancio del Senato (nota n. 18), il 50 per cento delle maggiori entrate, nel 2010, servirà a finanziare maggiori spese. Quindi, ci troviamo di fronte ad una ipotesi di aumenti di spesa nel triennio 2008‑2010. L'esatto opposto di quello che dichiara il ministro Tommaso Padoa-Schioppa. Questo quadro è reso ancora più drammatico dallo scenario macroeconomico che si prefigura nel prossimo triennio. Nel 2008 si prevede una crescita del PIL notevolmente rivista al ribasso: per cento previsto nel Documento di programmazione economico-finanziaria di giugno, la Commissione europea prevede una crescita dell'1,4 per cento e l'OCSE dell'1,3 L'indebitamento, senza l'approvazione dei decreti-legge nn. 81 e 159, varato qualche mese fa, sarebbe stato dell'1,8 e invece è stato rialzato al 2,5 per cento, grazie allo sperpero di due "tesoretti" del 2007. La spesa prevista dai due "tesoretti", derivanti da maggiori entrate per oltre 20 miliardi di euro, non è ristretta al solo 2007, ma per una parte si ripete nel 2008 e negli anni seguenti. Dove sta scritto che anche nei che anche nei prossimi anni avremo altri "tesoretti"? Anzi, una buona parte di queste entrate sono dovute ad una forte crescita del PIL nel 2007, che ha toccato il 2 per cento. Se nel 2008 si prevede una minore crescita della ricchezza di oltre mezzo punto percentuale di PIL, è ragionevole ritenere che ci saranno minori entrate; sicuramente non ci saranno i "tesoretti" che abbiamo conosciuto. Allora, come saranno pagate le maggiori spese decise nel 2007 anche per gli anni futuri? Mac'è di più. Il giudizio politico e morale di questo stato di cose sta nella ricaduta su pensionati e disoccupati. Infatti, l'aumento dell'inflazione, che è una tassa occulta che si scarica sui lavoratori a reddito fisso, è prevista al 2,3 per cento, secondol'ISTAT, ma tutti sanno che l'inflazione reale è pari al doppio di quella dichiarata dall'ISTAT. Ebbene, l'aumento di gas, luce ed acqua, l'aumento del gasolio e della benzina, su cui pesano le accise, determineranno paradossalmente un aumento delle entrate per Stato e Regioni. Come dire: piove sul bagnato. Quegli aumenti di qualche decina di euro per incapienti e pensionati saranno tutti assorbiti dall'aumento del costo della vita e quindi dall'inflazione. Senza trascurare che ci sarà a chi è andata peggio, perché eventuali benefici fiscali della prima ora sono stati riassorbiti dalle addizionali IRPEF di Regioni e Comuni. mi soffermo, per carità di Patria, su quelli ai quali è andata ancora peggio: mi riferisco ai redditi falcidiati sin dalla prima ora, cioè quelli sopra i 25.000 euro. Lariduzione del potere di acquisto di salari e stipendi per il 2008, insieme ad una riduzione della crescita del PIL che si attesta sotto l'1,4 per cento, significa rallentamento dell'occupazione e minori consumi interni. Posto che l'*ex**port* italiano, con il cambio euro-dollaro a 1.50, sarà fortemente ridimensionato nell'area del commercio dominata dal dollaro e che i capitali in euro voleranno verso investimenti a buon mercato dell'area dollaro, ben si comprende come il 2008 sarà un anno drammatico e a tinte fosche. Segli italiani non arrivavano alla quarta settimana del mese, immaginatevi se riusciranno a fare la terza. Soprattutto perché, con le minori entrate strutturali che vi saranno a legislazione vigente, non si potrà favorire una maggiore spesa pubblica per rilanciare i consumi interni. Anzi, per pagare le spese triennali o pluriennali che sono state fatte nell'anno dei "tesoretti", ci vorranno più entrate. Si pensi ai 10 miliardi di euro che serviranno nei prossimi dieci anni per pagare la pensione ai cinquantottenni prevista dalla riforma del *welfare*. L'unica strada è quella del taglio delle spese. Finora però tale strada è stata impraticabile. Allora? Che fare, amici del centro-sinistra? Questo Governo non è in grado di tagliare le spese, nemmeno quelle inutili o improduttive. Lo si è visto con i risultati conseguenti alla denuncia del libro verde sulla spesa pubblica: nessuna riforma nei meccanismi della spesa inefficiente è stata fatta. Questo Governo Prodi, però, non ha più la possibilità di aumentare le tasse neanche di un euro perché il Paese è ormai allo stremo. Quindi, niente tasse, niente tagli di spesa. Questo è il dilemma che abbiamo di fronte. Ora, è a tutti evidente che il Governo Prodi è a fine corsa. Non è più in grado di governare l'Italia perché ha troppe contraddizioni interne, sia di natura politica e sociale che di natura economica e di carattere etico. Questa amara constatazione ci porta ad un'altra constatazione ancora più amara: che questo Governo non ha alternative. Un Governo cade quando ne è pronto un altro, ma un altro non c'è, anche perché non c'è più nemmeno quello dell'incantesimo, cioè quello di Berlusconi, stante la fine della Casa delle Libertà voluta dallo stesso Berlusconi.

Se l'Italia si è paralizzata tra Prodi e Berlusconi, è altrettanto vero che solo con un passo indietro di tutt'e due, per il bene dell'Italia, si può immaginare un Governo alternativo a quello di Prodi e a quello di Berlusconi. Finché l'Italia rimane schiacciata tra Prodi e Berlusconi, gli italiani saranno sempre più poveri. Bisogna uscire da questo incantesimo o, meglio, da questa condanna storica, per restituire all'Italia un Governo libero e democratico. Noi dell'UDC avevamo indicato la strada di una riforma elettorale che superasse il vincolo delle coalizioni populiste ed elettorali per lasciare il posto alle coalizioni programmatiche e parlamentari. Anche questa strada è stata occupata con forza dall'asse Veltroni-Berlusconi, che rinnova il bipolarismo leaderistico Prodi-Berlusconi nella variante Veltroni-Berlusconi, che è la stessa cosa dei dodici anni trascorsi, senza che l'Italia abbia risolto uno solo dei suoi storici problemi strutturali. Italiani, aprite gli occhi. Lo voglio dire attraverso questo microfono: la politica che serve all'Italia non è quella del bipolarismo mediatico e muscolare, che ci propinano i sette telegiornali di Mediaset e RAI ogni sera. C'è bisogno di un'altra politica, quella delle riforme: dell'efficienza dei mercati; delle liberalizzazioni dei servizi pubblici locali e nazionali; dell'apertura delle professioni; di una scuola del merito; di una giustizia che funzioni; di banche meno esose e meno usuraie; di infrastrutture materiali ed immateriali efficienti e meno costose; di sicurezza sociale e personale; di flessibilità nel mercato del lavoro che non diventi precariato; di un fisco meno patrigno e più amico dei contribuenti; di più ricerca e meno assistenza pelosa per le aziende che vogliono competere; di chi sa scegliere il nucleare senza rinunciare alle energie rinnovabili alternative. È un'Italia diversa, moderna, efficiente, solidale quella che sogniamo. È l'Italia che rispetta la persona, che sa riconoscere la propria identità nazionale, che sa accogliere e ascoltare senza rinunciare a se stessa e a decidere. È un'Italia diversa da quella che abbiamo conosciuto in questi ultimi dodici anni. L'UDC voterà contro questo Governo, contro questo bilancio e contro la finanziaria che stiamo esaminando, perché rappresentano l'opposto dell'Italia che vogliamo. Signor Presidente, non è questo certo il clima di un grande confronto politico; tutti sappiamo il giorno e l'ora in cui si finirà con l'approvazione

Il giudizio è quello di una finanziaria che è migliore di quella dell'anno precedente perché non poteva essere peggiore, ma che è inadeguata ad affrontare i problemi del Paese. Vi ringrazio per l'applauso, ma non sarete d'accordo su come si conclude tutta la questione. PALMA *(FI)*. Aggiungerò di più per ringraziarvi di questo sostegno *bipartisan*, che è cosa diversa dal Veltroni-Berlusconi. In sostanza, nelle discussioni che abbiamo sviluppato all'interno del nostro movimento, che non interesseranno sicuramente i nostri un giudizio fortemente critico sulle attuali competenze acquisite dai partiti: strapotere e mancanza di democrazia all'interno dei partiti; zone grigie sui finanziamenti e sulle nomine dei dirigenti e dei parlamentari. Il guaio è che ci troviamo di fronte alla proposta di legge elettorale Veltroni-Berlusconi che peggiora la situazione. L'immagine che abbiamo visto è quella del Castello estense di Ferrara, che fu costruito - come è notorio - non contro l'invasione delle altre realtà che contornavano il Ducato degli Estensi, ma per difendere i signori di Ferrara dal proprio popolo:

a qualche forza politica che volesse stare fuori dal coro e da questo teatrino della politica e che potrebbe rappresentare un rischio. Un rischio per chi? per chi? Per quei soggetti finanziari, più che imprenditoriali, che da un lato fanno i padrini del nuovo Partito Democratico, ma che poi troviamo nelle banche, nei servizi pubblici, pubblici, nelle aziende di Stato acquistate a prezzo stracciato, nell'editoria, nella realizzazione dei turbogas e degli inceneritori, ossia quei grandi finanzieri che vivono sul danaro pubblico italiano, ma che dai loro giornali - dal «Corriere della Sera», «La Stampa» e «la Repubblica» - da anni ci pongono il problema che il bipolarismo non va più bene, che bisogna andare al bipartitismo e che i due partiti devono essere talmente simili e dipendenti dal loro sistema di potere che, che, vinca Tizio o vinca Caio, sono comunque garantiti e continueranno a fare il bello e il cattivo tempo in questo Paese. Per tornare invece alla Costituzione, la quale prevede che sia libera l'associazione in partiti nel nostro Paese, che assomiglia purtroppo sempre più ad un regime più che ad un sistema democratico (basti vedere come, oltre alla stampa, vengono usati i mezzi televisivi), poniamo l'esigenza che ci sia un proporzionale. Quanti sono i seggi? Il numero dei votanti rapportato al numero dei seggi fa la quota per avere un seggio. Tutti i trucchi che si stanno studiando adesso per tradire il voto degli elettori e portarlo, assieme al finanziamento pubblico, o verso Berlusconi o verso Veltroni oppure per far passare gli eventuali alleati sotto le forche caudine dell'ubbidienza tacita, sono forme antidemocratiche.

bastava parlare di un milione in più per gli invalidi, un milione in più per "vita indipendente", un miliardo per le povertà, che i soldi non c'erano.

Siamo ancora ai mille rivoli per accontentare chi più, chi meno. C'è un'aria un po' troppo preelettorale all'interno di questa legge finanziaria. Non so se il Governo Prodi sia a favore dell'eutanasia, nonostante la sua componente *teocon*, e cioè se sia consenziente alla fine o se sia invece un assassinio quello che sta per essere preparato con la proposta della legge elettorale e con i mal di pancia che qua e là si avvertono dopo il *big bang* del Partito Democratico. Sta di certo, però, che continuare a non governare e a non fare le scelte è il modo migliore per far finire questo Governo, a cui non siamo particolarmente affezionati; qualora emerga una proposta politica, un *micron* migliore dell'attuale Governo, siamo pronti a cambiare posizione politica. Per ora vorremmo evitare la caduta di questo Governo perché non sappiamo dove si andrà a sbattere. Uno dei freni era la questione della guerra. Apprendiamo dal recente viaggio in America del Presidente della

Alla faccia della nostra sinistra in naftalina, che è pronta a credere a tutto quello che D'Alema racconta, perché D'Alema è il «miglior figo del bigoncio» ed è molto intelligente. altro elemento del viaggio americano che stupisce, perché il presidente Napolitano è di Napoli,

Ma non si sono accorti che dal 1995 in America gli inceneritori non li fanno più? Qui li chiamiamo termovalorizzatori, ma non solo: diciamo che non ci sono soldi, ma ad ENI, ad

ci sono i morti, le malattie invalidanti che sono frutto delle nanopolveri. Ci dicono che le nanopolveri non ci sono.

Si riconoscono i danni da nanopolveri, ma non si vuole ragionare sul fatto che le centrali a turbogas e gli inceneritori creano tonnellate di nanopolveri e producono morti e malattie invalidanti che ricadono sul Sistema sanitario nazionale. Pochi guadagnano molti soldi, molti ci rimettono in salute, ma paga lo Stato. *(AN)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, già il senatore Vegas questa mattina, nel presentare la relazione di minoranza nell'ambito della Commissione bilancio, ha avuto modo di

vero e proprio assalto alla diligenza. È un modo vergognoso per due ragioni, signor Presidente. Prima Prima di tutto, il Governo, nello scrivere il maxiemendamento sul quale ha chiesto la fiducia, accorpando in tre capitoli la legge finanziaria - il bilancio ovviamente è la conseguenza contabile e numerica di tutto questo si è basato su un presupposto francamente offensivo e cioè che, a partire dalla propria maggioranza, per arrivare ai membri del Parlamento di opposizione, per giungere fino ai cittadini italiani, siano tutti sciocchi e cretini e non in grado di leggere un testo che, seppur in giuridichese, è pur sempre scritto in lingua italiana. Da questo punto è vergognoso che il Governo chieda la fiducia su quel tipo di testo. Il collega Vegas stamattina ha fatto esempi clamorosi. Si chiede la fiducia - mi limito ad uno solo, il più esilarante

per ogni 6 kilowatt di energia elettrica consumata. Risparmio a lei, signor Presidente, ed ai colleghi, ulteriori esempi di questo tipo che però già il collega Vegas ha avuto modo di

ringraziando ovviamente per tradizione il Governo che nel testo che ci è pervenuto dalla Camera rileva in neretto le modifiche, per cui è più facile vedere le nefandezze scritte - ne abbiamo rilevate

ed è più serio in termini di responsabilità economico-finanziaria e quindi politica e di responsabilità istituzionale. Signor Presidente, il ragionamento purtroppo proviene da lontano, sin dal primo momento in cui questo Governo ha fatto sentire i propri vagiti dopo la nascita.

ma io, per essere più aderente all'italiano risciacquato in Arno, elenco le sette bugie capitali, quasi i sette peccati capitali, che il Governo ed il Ministro dell'economia hanno detto al Parlamento. Signor Presidente, cari colleghi, indipendentemente dalla maggioranza o dall'opposizione, è chiaro che il Ministro dell'economia ha ripetutamente mentito al Parlamento, reiterando menzogne e bugie. Vado per titoli, signor Presidente. Cito per primo il caso Alitalia: all'inizio di dicembre dell'anno scorso si annuncia una privatizzazione della compagnia con una procedura cervellotica che negli ambienti finanziari di Londra, di Francoforte, di New York è stata da tutti considerata inaccettabile per un Paese civile. È una procedura che si basa su chi vuole mandare lettere di intenti al Ministero dell'economia, che mette alla fine del processo, immaginato per giugno di quest'anno, la proposta di piano industriale di chi fosse interessato alla compagnia Alitalia. di febbraio e marzo, rispondendo con la consueta sollecitudine il Ministro dell'economia ha svolto un'audizione alle Commissioni congiunte bilancio e finanze della Camera e del Senato, rispondendo ad una mia personale richiesta urgente effettuata il 18 dicembre 2006, due mesi e mezzo prima. In quella audizione ha ripetuto la menzogna e ci siamo trovati negli ultimi giorni a celebrare il massimo - non saprei dire - se della ignoranza o dell'arroganza: probabilmente delle due cose insieme, che è la peggiore miscela che possa mai determinarsi, non solo in politica ma in ogni campo della vita civile.

(non per conto di se stesso o di altri azionisti di maggioranza occulti di questo Governo e che non siedono nelle Aule parlamentari),

avendo perso l'occasione che tutti gli analisti da anni denunciano. Infatti, una compagnia come l'Alitalia, decotta da anni sul piano delle condizioni economico-finanziarie, ha solo un'opportunità da offrire eventualmente a *partner* internazionali: quella di divenire la base strategica in Italia, in Europa e nel Mediterraneo per qualche compagnia del Nord-America o dell'Asia. Questo è il valore dell'Alitalia. Seconda bugia: il Ministro dell'economia ci ha detto che lui poteva cacciare un consigliere di amministrazione della RAI; mi sembra che qualche giudice abbia detto che invece non poteva farlo. Terza bugia: il Ministro dell'economia,

che a un anno dai fatti che lui denunciava sentiva doveroso rimuoverlo e, contemporaneamente, proporlo come consigliere di Stato. merito a questo nei giorni recenti qualche giudice fortunatamente e ancora per la correttezza istituzionale e democratica dell'Italia ha detto che non poteva farlo. quarta bugia riguarda più il merito del ruolo specifico del Ministro dell'economia e delle finanze. I casi che ho ricordato riguardano il Ministero dell'economia ma è chiaro che la madre di tutte la responsabilità del Ministro dell'economia è la politica economica. Ebbene, la quarta bugia questo Governo l'ha detta sempre nelle Aule parlamentari all'inizio del suo mandato, quando è venuto a raccontare che era costretto a fare una maximanovra da 45 miliardi di euro di maggiori tasse perché la situazione era assolutamente tragica, tragica, sull'orlo del tracollo e del collasso, peggiore di quella del 1992, che portò alla nota crisi della lira.

Ha ragione il collega Rossi: questa finanziaria è un po' migliore solo perché non poteva essercene una peggiore; ma è vergognosa, collega Rossi, perché ha caricato sulle spalle dei lavoratori italiani 45 miliardi di euro di tasse in più, non per riparare ad una situazione di squilibrio finanziario ma per creare una marmellata da distribuire in mille rivoli

dopo parecchie insistenze, il collega Visco venne in Commissione bilancio e poi in Aula e, l'11 dicembre dell'anno scorso, portò la tabella della verità. se quella era la tabella della verità sull'andamento del gettito del 2006 che incorporava i dati dell'acconto di novembre (quindi i preconsuntivi più solidi); se quella che Visco ha portato in quest'Aula era la tavola della verità, quello che ha detto il Ministro dell'economia era la più clamorosa delle menzogne, tanto che lo scorso anno

(quello dell'IVA sulle automobili e il debito della TAV), e li ha contabilizzati nel *deficit* pubblico, perché altrimenti

del bilancio 2007, quel gettito palesemente sottostimato è stato fatto emergere a pezzi a marzo, a giugno, a luglio, a fine luglio, a fine agosto, ai primi di settembre e attraverso ben sei tesoretti successivi, definiti come lotta all'evasione fiscale. Anzi, poiché probabilmente ha più frequentazioni anglosassoni che con il popolo italiano, il Ministro dell'economia ha avuto il pudore di scrivere formalmente nei suoi documenti ufficiali che si tratta di *tax compliance*:

nascosto in precedenza e fatto emergere a pezzi, il Governo ha ritenuto che era giunto il momento di spenderlo. Più volte ci siamo sentiti dire

Ebbene, si spendono 7 miliardi nel decreto di luglio (primo decreto tesoretto); si spendono 8 miliardi nel decreto del 1° ottobre (secondo tesoretto);

E la sesta bugia è derivata da un semplice fatto: abbiamo l'extragettito, lo possiamo spendere.

di 1,35. Il Governo si è accorto che questi dati oggi sono radicalmente mutati? La sua colpa non consiste nel cambiamento di questi dati e di questo scenario, ma è una colpa politica e istituzionale non prenderne atto.

Sulla base dei dati ufficiali del Governo, in assenza di queste manovre che ha fatto e ci propone (e cioè i 31 miliardi di spesa in più, introdotti da luglio ad oggi,

la stabilizzazione dei precari nelle pubbliche amministrazioni e - collateralmente, nel provvedimento sul *welfare*

con il pericolo di una forte frenata dell'economia, si sta facendo correre al Paese, qualunque sia il Governo che ci sarà ad aprile o maggio, di essere richiamato all'ordine dall'Unione Europea per una manovra correttiva in corso d'anno, nel momento in cui l'economia starà già frenando e frenando

non dobbiamo sorvolare sulle critiche che sono state sollevate, anche nel dibattito che si è sviluppato in

nei ruoli di Governo o alla guida delle Commissioni - ad essere più rigorosi nello stabilire barriere alle norme che

nel modo migliore e più virtuoso che la situazione suggeriva, vale a dire se l'abbiamo utilizzato, per esempio, prevalentemente per ridurre il debito o per il miglioramento dell'incidenza del fabbisogno. Da questo punto di vista, penso che nell'analizzare il risultato finale di questa operazione, soprattutto da parte dell'opposizione, è difficile non tener conto di quale sia stato il comportamento di chi ha governato per cinque anni in una condizione dettata dai caratteri macroeconomici di allora e quale sia stata la differenza tra allora ed oggi. Ieri, vale a dire nella passata legislatura, di una crescita dell'economia sostanzialmente zero, quale quella che si è registrata nel corso di quegli anni) si è avventurato in una riduzione della pressione fiscale che ha finito per interessare prevalentemente, per così dire, settori di contribuenti dai gli scarsissimi risultati che si sono registrati perché ciò non ha per niente provocato una crescita della domanda interna e quindi una ripresa dell'economia e si è completamente mangiato l'avanzo di amministrazione ricevuto in eredità dal precedente Noi, in presenza di una situazione che ha rivisto una ripresa e sostanzialmente una economia in crescita, abbiamo deciso prevalentemente di occuparci delle fasce più deboli e quindi abbiamo rivolto la nostra attenzione

un'attenzione esattamente opposta a quella che il Governo precedente aveva rivolto verso le fasce medio-alte. Ci siamo preoccupati di riprendere una politica per la casa, che era assente da oltre dieci anni in questo Paese, in particolare rivolgendoci al settore degli affitti, e quindi alle famiglie famiglie monoreddito, per aiutarle a sostenere la spesa dell'affitto di casa e abbiamo avviato una fase di riduzione della pressione fiscale che ha interessato prevalentemente le imprese, con la finanziaria dell'anno scorso, che è proseguita quest'anno, facendo le operazioni che conosciamo e che sono state anche ricordate. Si tratta, quindi, sostanzialmente di due filosofie di approccio completamente opposte. Abbiamo pensato di mettere i conti a posto, sulla base di una maggiore entrata che era determinata da una maggiore crescita ci siamo preoccupati di ripristinare l'avanzo, di cominciare a riaggredire il debito e di dare qualcosa alle fasce più deboli della nostra società. Allora, il vero punto controverso ancora presente nella nostra discussione, e che non trova soluzione, è la ragione per la quale noi cresciamo meno degli altri Paesi dell'euro: mediamente mezzo punto, quando non oltre, meno degli altri. C'è, quindi, un problema di competitività del nostro sistema produttivo, che penso il collega Baldassarri non vorrà imputare esclusivamente a questi primi due anni di Governo del centro-sinistra, perché si tratta di fattori strutturali che vengono da molto lontano. Vorrei qui ricordare, sempre per equità del nostro confronto dialettico, che nei cinque anni di Governo del centro-destra nulla è stato fatto per migliorare la competitività del sistema o in termini sistema o in termini di liberalizzazioni dell'economia del Paese. Nulla è stato fatto per l'Alitalia, che si trova in questa situazione anche perché durante quei cinque anni di Governo non si è prestata assolutamente attenzione alla disastrosa situazione dei conti della compagnia, che noi abbiamo evidentemente ereditato e a cui cerchiamo oggi con difficoltà di trovare una soluzione. il terreno sul quale dobbiamo impegnarci di più è quello della competitività del sistema; l'altro è quello del miglioramento della nostra capacità di ridurre la spesa. Ma anche qui avendo un'attenzione: la spesa non può essere ridotta in modo general-generico, bisogna capire dove occorra ridurre. Per esempio, sicuramente non dobbiamo ridurre la spesa sanitaria, anche per gli ultimi elementi che ci sono stati forniti al riguardo sul rapporto tra il servizio che offriamo e quello che spendiamo per realizzarlo rispetto ad altri Paesi. Non possiamo ridurre la spesa nella scuola e nell'istruzione. Non possiamo ridurre la spesa nella ricerca, anzi, possibilmente la dobbiamo incrementare. C'è evidentemente un tema della spesa nell'apparato della pubblica amministrazione che rimane il cuore dei nostri problemi, per il quale nei cinque anni di Governo del centro-destra non è stato fatto assolutamente niente; quindi, da questo punto di vista non possiamo ricevere lezioni a a proposito della nostra scarsa capacità di ridurre la spesa. Ci stiamo applicando, stiamo cercando di farlo in maniera selezionata e devo dire che la doppia lettura fin qui registrata (questa è la terza) mette in evidenza che qualche miglioramento il Parlamento questa volta ha fatto anche anche al riguardo. Si tratta di proseguire su una linea che abbiamo tenuto con queste due finanziarie, che ci consente di agire concretamente nella direzione che conferma una coerenza nel rigore, nel rispetto dei conti, quindi dei parametri della finanza pubblica, che conferma un'azione di equità nella riduzione della pressione fiscale e non una generica riduzione della pressione fiscale senza che questa comporti una selezione del modo in cui bisogna farla, una lotta all'evasione fiscale che nessuno qui ha voluto sottolineare essere uno dei titoli che fa aumentare le entrate fiscali dell'ultimo periodo, una riduzione del peso del debito. Oggi su tutti i giornali la Spagna domina perché ha superato l'Italia in termini di ricchezza *pro capite*; è sicuramente un dato negativo, perché è sempre meglio competere crescendo. Questa volta siamo stati superati da un Paese che - bisogna ricordarlo - non è grande come il nostro; anche la dimensione del Paese va tenuta presente quando si analizzano i dati, ma se si osserva quali sono i fattori principali che determinano la crescita della Spagna, c'è la fotografia esatta di quanto dicevo prima: un Paese che ha un peso di aziende pubbliche enorme rispetto all'altro, un Paese che ha un grandissimo numero di aziende private, e tutto ciò ovviamente non è solo il frutto di questi due anni di Governo, ma anche del fatto che nei cinque anni del Governo precedente nulla si è fatto per migliorare le condizioni generali. Dalla Spagna occorre cogliere non solo gli indicatori economici, ma anche e questo può essere tema di questi giorni in cui discutiamo di riforme istituzionali e di politica - gli aspetti politici; sicuramente in quel successo c'è anche il fatto che due forze politiche alternative fra di loro per il Governo sono però unite nell'interesse del Paese

una sfida sul terreno della competizione a migliorare il nostro sistema, ma anche una sfida sul terreno politico che forse faremmo bene a cogliere in questi giorni di discussione su riforme istituzionali e su legge elettorale. *(Applausi dal

vorrei aprire il mio intervento sulla manovra finanziaria 2008, che torna al Senato per la terza lettura, fornendo qualche dato numerico assai eloquente, a dimostrazione della chiarissima bontà del provvedimento, che verrà definitivamente licenziato nelle prossime ore, e dell'ottimo lavoro

sento ripetutamente parlare di falso in bilancio, di assalto alla diligenza; mi sembra di ricordare un famoso film di Massimo Troisi e Roberto

anche perché nella diligenza che noi abbiamo ereditato non c'era nulla; anzi, l'abbiamo dovuta rimettere in sesto per farle riprendere il giusto cammino. Infatti, dopo quattro anni consecutivi di sforamento dei parametri europei, nel 2007 il disavanzo pubblico è finalmente rientrato sotto la soglia del 3 per cento del PIL, su un valore del 2,4 Questo è senz'altro il migliore risultato da sette anni a questa parte. Rispetto a poco più di un anno fa, le finanze pubbliche italiane sono pienamente tornate sotto controllo. Questi risultati sono frutto di un serio e costante lavoro di contrasto all'evasione fiscale, che ha permesso un buon recupero di gettito fiscale e un nuovo controllo sulle spese, frenando l'andamento pericoloso in aumento, con un'operazione fondamentale di riqualificazione della stessa spesa pubblica. Si è proceduto poi ad una più equa redistribuzione della ricchezza, rispondendo innanzitutto alla necessità di sostenere i redditi dei ceti sociali più disagiati e di investire sul futuro, concentrando più risorse a favore dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese. Dunque, voglio ripeterlo, questa è una buona finanziaria e lo è per gli effetti immediati e tangibili che avrà, ad esempio, su famiglie e imprese. Per le famiglie, cito solo qualche solo qualche dato significativo. Il 40 per cento dei 43 milioni di persone che vivono in case di proprietà non pagherà più l'ICI. La restante parte avrà uno sgravio fino ad un massimo di 200 euro; è prevista l'esclusione dal beneficio per chi possiede ville, castelli o case di lusso. Ancora, è prevista un'importante novità per 2.800.000 persone che vivono in affitto, i cui costi negli ultimi anni sono lievitati in maniera preoccupante. Tali soggetti avranno una detrazione IRPEF da 150 a 300 euro, che aumenta per i giovani tra i venti e i trenta anni e che andranno a vivere da soli. Altra fondamentale misura, fortemente voluta dall'UDEUR, è quella che intende offrire un sostegno alle famiglie e alle persone che hanno sottoscritto un mutuo per l'acquisto della prima casa e che per diversi motivi possono trovarsi in situazioni di insolvenza. I dati economici diffusi dagli istituti bancari italiani testimoniano difficoltà crescenti per quanto concerne il pagamento delle rate del mutuo per la prima casa, un fenomeno sicuramente aggravato dalle variazioni al rialzo del costo generale del denaro, determinate dalla Banca centrale europea, che gravano soprattutto su chi ha acceso un mutuo a tasso variabile. Secondo i dati diffusi, dal 2002 al 2006, le famiglie che si trovano in difficoltà per quanto concerne il pagamento dei mutui sono passate da 356.000 a 408.000 e, solo nel corso del 2006, tali cifre hanno registrato un 5 per Riteniamo che l'importanza dell'abitazione, bene primario per ciascuno di noi e ancora più per le giovani coppie che costruiscono intorno alla prima casa buona parte del loro futuro, debba ricevere adeguate attenzioni e tutela da parte del legislatore. è stata inserita la misura che istituisce il Fondo di solidarietà per i mutui destinati all'acquisto della prima casa. Il Fondo interviene assumendosi il costo delle procedure per lo slittamento delle rate, che è possibile per non più di due volte e fino ad un massimo di diciotto mesi complessivi. Passo ora alle disposizioni relative alle imprese. Per i piccoli imprenditori - stimati in circa un milione - con un fatturato annuo sotto i 30.000 euro lordi, è previsto l'esonero del versamento dell'IRES e dell'IRAP e pagheranno solo a *forfait* un'aliquota del 20 per cento. Vorrei infine fare menzione di un'importante modifica contenuta in uno dei maxiemendamenti del Governo, presentati alla Camera. Si tratta dell'innalzamento del tetto del 5 per mille da 100 a 380 milioni, un investimento fondamentale per ricerca e terzo settore, che ha comportato un'impegnativa ricerca della copertura finanziaria, in tempi di risanamento. Concludo osservando che una buona legge, come la finanziaria e l'intera manovra 2008, non può essere considerata la panacea di tutti i mali del Paese. Certamente, però,

Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, ci apprestiamo a votare una finanziaria - e io lo farò convintamente - perché contiene molti provvedimenti a favore della tutela dell'ambiente, anche se per onestà bisogna dire che questa stessa legge finanziaria non è adeguata

nella scorsa finanziaria del 2007 e quindi procedono in quest'inversione di tendenza molto netta rispetto ad una strada opposta che nei cinque anni precedenti il Governo di centro-destra aveva perseguito,

di seguire anche in questo Paese la strada che in altri Paesi europei, come la Germania e la Spagna in particolare, è stata seguita per il rilancio e la grande diffusione di energie rinnovabili, quali l'eolico e il solare.

del registro nazionale dei serbatoi di carbonio che servirà a misurare l'effetto positivo che le foreste nel nostro Paese possono avere nel combattere l'effetto serra. serra. Ricordo poi la possibilità che si dà ai Comuni di diminuire l'ICI per quegli edifici in cui vengono utilizzati i pannelli solari e comunque le fonti di energia rinnovabile,

soltanto il divieto di vendita di apparecchi elettrodomestici e lampadine ad alto consumo energetico nel periodo dal 2010 al 2011, ma il combinato disposto del divieto di vendita dal 2010 senza aver inserito un incentivo alla rottamazione e, quindi, aver favorito i nuovi e più efficienti apparecchi - determinerà il rischio molto concreto che nei prossimi due anni il nostro mercato possa essere invaso da apparecchi sotto costo di bassissima efficienza. È del tutto evidente che, se dal 2010 e dal 2011 non si possono vendere e non c'è un adeguato incentivo per quelli ad alta efficienza energetica, si potrebbe persino ottenere il risultato opposto. Il problema strutturale che questa finanziaria non affronta - e che, quindi, la rende inadeguata rispetto al problema globale cui facevo è la questione che né nel settore dell'energia, né soprattutto in quello dei trasporti, si fanno quelle scelte, radicali da questo punto di vista e necessariamente diverse dal tran tran quotidiano, che servirebbero a rispondere al problema dei cambiamenti climatici. Altrimenti, non si spiegherebbe perché continuiamo a finanziare, magari a pioggia, con tanti piccoli interventi, una variante da una parte, un passante dall'altra, tante nuove strade ed autostrade e non si riescono a trovare i soldi per avere dei treni per i pendolari degni di un Paese civile. Non si spiegherebbe, inoltre, perché non si fanno quegli investimenti infrastrutturali e quelle grandi opere che renderebbero la rete ferroviaria italiana in grado di trasportare uomini, donne, e merci soprattutto, in maniera non dico rivoluzionaria, ma almeno pari a quello che succede in altri Paesi europei. Questo è il punto. D'altra parte, nel passaggio alla Camera, abbiamo assistito purtroppo ad alcuni provvedimenti che lasciano veramente con l'amaro in bocca. Non si potrebbe

è sempre stata in difficoltà e negletta e per cui noi dovremmo avere la responsabilità di aumentare i fondi. Alla fine, *in extremis*, si sono tolti quei 92 milioni di euro per dare un ennesimo sconto al sistema dell'autotrasporto che oggi è basato esclusivamente sui Tir, rinunciando, ad affrontare, una volta per tutte, la necessaria inversione di tendenza nel sistema di trasporto delle merci nel nostro Paese.

provvedimenti di settore che lasciano sorpresi e perplessi. Mi riferisco a quando, per esempio, si è voluta inserire in finanziaria l'ennesima proroga per lo smaltimento in discarica dei rifiuti tal quali si è voluta inserire, sempre in finanziaria, l'ennesima proroga che permette ai Comuni di non passare da tassa a tariffa, anche se questo sarebbe l'unico modo per aumentare davvero la raccolta differenziata e passare alla gestione integrata dei rifiuti. Quando si sceglie di concedere

passaggi fondamentali. Certo, molto ha a che vedere con la modalità con cui la legge di bilancio e quella finanziaria - è stato detto da molti colleghi e dal relatore

è davvero, da una parte, un'urgenza non più rinviabile ed una necessità da affrontare - altrimenti si va incontro a dei rischi enormi - e, dall'altra, un'opportunità per la modernizzazione del sistema nel suo complesso. [**Presidenza del

Volevo dare atto al collega Randazzo di aver a me e al collega Saro sostanzialmente confermato quanto già dichiarato agli organi di stampa, ossia di avere avuto con il presidente Berlusconi un colloquio assolutamente corretto in ordine al quale non aveva alcunché di cui lamentarsi né sotto il profilo etico, né sotto quello strettamente politico. Per il resto, Presidente, vorrei dire quanto segue. Il collega Randazzo mi ha detto di essere stato effettivamente sentito dai pubblici ministeri di Napoli due o tre giorni prima del voto sulla finanziaria. Mi chiedo se una tale attività, in assenza della rilevanza dei fatti sulla base delle stesse dichiarazioni del collega Randazzo, e principalmente in assenza di qualsivoglia tipo di urgenza, non sia oggettivamente da considerare come incidente sulla libertà di voto dei senatori in genere; ciò anche alla luce del fatto, signor Presidente, che già il collega Mancuso era stato oggetto di una denuncia - uso il termine evidentemente in modo improprio - della Commissione antimafia, presieduta dal senatore Centaro, nella precedente legislatura, legislatura, in virtù della quale era stato richiesto al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura di attivare le iniziative del caso. Aggiungo, signor Presidente, non per gettare una luce oscura su tutta la vicenda, ma oggettivamente per ripetere dei fatti, che trovo davvero singolare che il pubblico ministero di Napoli credo nella contestualità dell'esame del senatore Randazzo - si sia incontrato (così pare emergere da notizie di stampa) con il presidente Violante. A questo punto, mi chiedo con chi altri si sarà incontrato

Per il futuro, non sono interessato a passi indietro, in quanto - come mi pare risultare dalle voci insistenti che circolano negli ambienti istituzionali - il dottor Mancuso lascerà probabilmente la procura della Repubblica di Napoli

Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, dopo il passaggio sia al Senato che alla Camera, riteniamo che la manovra sia rimasta sostanzialmente inalterata nei suoi obiettivi principali, che sono quelli di ridimensionare il debito pubblico e non solo: accanto al risanamento dobbiamo pensare anche allo sviluppo e all'equità.

Sul fronte del risanamento, è vero che la manovra lorda - come ci ha ricordato il relatore - ha certamente registrato un incremento che l'ha portata dai circa 11 miliardi euro iniziali ai 15,5 miliardi di euro nel suo importo complessivo (il passaggio al Senato ha visto aumentare la manovra lorda di 1,9 miliardi e il passaggio alla Camera di 2,2 miliardi). Tuttavia, va sottolineato che il saldo netto da finanziare è stato migliorato nel corso dell'esame parlamentare

Le compensazioni reperite a copertura dei maggiori oneri, infatti, sono state in larghissima parte concentrate su ulteriori riduzioni di spesa, mantenendo pressoché inalterata la pressione fiscale, obbiettivo che la maggioranza si era data all'inizio del percorso della manovra.

che riduce in modo molto significativo l'aliquota IRES per le società di capitali. In proposito bisognerà appunto verificare se questo intervento non crei una disparità o piuttosto sia, come speriamo, un incentivo alla capitalizzazione delle imprese individuali e delle società di persone. normativo sicuramente va nella direzione di rafforzare, anche attraverso una maggiore trasparenza nel rapporto tra imprese - o contribuenti più in generale - e Stato, la capacità competitiva del Paese sotto il profilo di una riforma del sistema fiscale.

sull'addizionale comunale IRPEF, che dal 2008 vedremo applicata concretamente nel nostro Paese; una misura che chiamo federalista perché prevede che, attraverso l'assegnazione di un codice tributo, i nostri Comuni incasseranno direttamente l'addizionale comunale IRPEF prodotta e pagata sul loro territorio. Il presente disegno di legge avvia anche un ulteriore percorso federalista che è quello della regionalizzazione dell'IRAP, pienamente effettivo dal 2009.

che è stato fatto in passato, almeno nel recente passato. Sul piano federalista, devo dire che un passo indietro - e questo va riconosciuto, una critica in proposito va sollevata per essere autenticamente e convintamente federalisti - è stato compiuto a proposito dello

Accanto alla previsione di un aumento di 190 milioni di euro in finanziaria per il rinnovo e l'ammodernamento dei mezzi e degli aeromobili delle forze di Polizia e dei Vigili del fuoco - una misura che segna

Interessante - vado avanti con altri esempi concreti - anche la norma che prevede un incentivo ai proprietari di edifici in centri storici a provvedere al loro risanamento, riqualificazione e restauro. Credo che combattere

ai titolari di edifici situati nei centri storici fino ad importi di 300.000 euro con interessi totalmente a carico dello Stato è una norma particolarmente significativa. Significativa è anche l'introduzione nella legislazione nazionale di un principio perequativo nell'edilizia residenziale, volto a favorire la realizzazione di edilizia sociale e di servizi alla persona.

numerosi contenziosi. Questi sono solo alcuni esempi della concretezza di questa finanziaria. Cito

non può che passare finalmente attraverso una più coraggiosa iniziativa in sede riformatrice. Mi pare che nella finanziaria si concentrino tutte le attese ed i tentativi di legiferare e di dare soluzione ai problemi di un Paese. Non può essere la finanziaria lo strumento che dà risposta a tutte le gravi questioni questioni che il Paese ha di fronte a sé per evitare il declino e riprendere un sentiero stabile di crescita. Su versante delle riforme stiamo facendo ancora poco. Ci sono difficoltà anche di tipo politico che non sono solo della maggioranza; c'è anche la difficoltà di collaborazione su questi temi,

nella sua parte iniziale, cioè la questione salariale. La questione di ridare potere d'acquisto alle nostre famiglie e di fare riprendere la crescita ed i consumi. Da questa finanziaria, ormai già alle nostre spalle, dobbiamo quindi ripartire con la consapevolezza che il nostro compito è quello di aggredire in modo più efficace, attraverso riforme importanti, la spesa pubblica non tanto nel senso di una sua riduzione, che auspichiamo ma che crediamo difficile nelle condizioni date, ma nella direzione di una vera, seria ed efficace sua riqualificazione: spendere bene le risorse che i cittadini ci mettono a disposizione con la fiscalità,

Signor Presidente, il passaggio alla Camera dei provvedimenti finanziari ed il loro ritorno al Senato non ha mutato il giudizio che ho su questa manovra economica. Lo sintetizzo così: in primo luogo, dissento profondamente dal fatto che dal 2007 alle imprese, alle banche e alle assicurazioni è stato garantito la più grande tassazione della storia: 7 miliardi ogni anno. Nel 2008 sono confermati e ad essi si aggiunge anche l'abbattimento di IRES e IRAP. Ma in finanziaria, mi pare ci siano tanti altri sgravi, facilitazioni ed incentivi, sempre per le imprese per centinaia di milioni. Al contrario, non vedo le misure di tassazione delle rendite finanziarie e tanto meno un forte intervento a favore dei salari, ormai ridotti alla fame. Si rinvia continuamente. In sede di dibattito in prima sessione mi è stato detto, respingendo i miei emendamenti, che puntavano a dare ai giovani un po' di sicurezza con il salario sociale ed a restituire ai lavoratori il *fiscal drag*: «Vedremo, se ci sarà un tesoretto prossimo forse interverremo». Ma così siamo ben lontani dal risarcimento sociale promesso. Proprio in questi giorni molti lavoratori e lavoratrici mi hanno testimoniato di aver ricevuto stipendi e tredicesime più sottili e leggere. Dove sono finiti i problemi di sopravvivenza delle famiglie? Dov'è finita la quarta settimana? Si parla dell'aumento dei prezzi, certamente, è giusto perché gravissimo, pesa fortemente non solo sulla quarta ma anche sulla terza settimana, però era ora il tempo di intervenire, non di promettere qualcosa per domani. È curioso che le organizzazioni sindacali chiedano la restituzione del *fiscal drag* a gennaio, guarda caso, guarda caso, a manovra finanziaria chiusa. E già molti mettono le mani avanti sul prossimo tesoretto, se ci sarà, a partire dal Ministro dell'economia, che si affretta a dire che, in primo luogo, rimane il problema del risanamento, da una Corte dei conti che dice che già il precedente tesoretto doveva essere utilizzato solo per il risanamento, e

Altro che quarta settimana. E che tempistica queste uscite, proprio nel momento in cui 7 milioni di lavoratrici e lavoratori ancora stanno lottando, mobilitandosi per rinnovare il loro contratto di lavoro.

Terzo elemento di non condivisione, che è forse quello che più di tutti mi appassiona e mi rende anche molto preoccupato.

per le vittime dell'amianto. È incredibile una situazione di questo genere. Per tutte queste ragioni, collegate anche al giudizio che darò sul Protocollo del *welfare,* il mio giudizio ed anche il mio voto sono negativi.

Addirittura, con un attacco diretto da Bruxelles, veniva evidenziato come avessimo avuto per tutta la scorsa legislatura, ad eccezione di un anno, un *deficit* superiore al 3 per cento del PIL. Il debito pubblico aveva ripreso a salire dopo una decennio, l'avanzo primario era stato azzerato, la spesa primaria corrente era cresciuta di 2,4 punti di PIL durante i cinque anni precedenti, raggiungendo il livello *record* del 40 per cento del PIL. Neanche nei primi anni Novanta la spesa primaria corrente aveva toccato tali livelli. Queste erano le condizioni quando il Governo si è insediato: vi era un'emergenza che occorreva affrontare in maniera risoluta per non penalizzare ulteriormente le giovani generazioni e dare prospettive di stabilità all'intera economia. a distanza di meno di due anni, il *deficit* pubblico, non solo, è stato riportato ampiamente sotto la soglia del Trattato di Maastricht, ma tutto ciò è accaduto senza ricorrere a misure *una tantum*; le stesse misure *una tantum* che - è bene sottolinearlo - nella scorsa legislatura sono state utilizzate con inedita larghezza per un importo complessivo di ben 64 miliardi di euro. Il debito pubblico è ora in discesa, l'avanzo primario, un tempo azzerato, ora viene ricostituito. Ciò è il risultato di più fattori: in primo luogo una crescita maggiore e più sostenuta rispetto al passato recente, ma anche soprattutto un ritorno alla legalità e alla disciplina da parte dei contribuenti indotto dalle nuove e più rigorose politiche fiscali del Governo. La legge finanziaria dello scorso anno e quella oggi in discussione vanno guardate in prospettiva; esse vanno inserite nella realtà dei conti pubblici che abbiamo dovuto affrontare e degli obiettivi che si impongono nei prossimi anni. Non daremo nessun futuro ai giovani se non abbatteremo il debito e se non libereremo ricorse per maggiori e migliori beni e servizi pubblici: migliori strade, miglior insegnamento, migliore ricerca, maggior sicurezza, giustizia più rapida e migliori mezzi di trasporto. Il profilo originario di rigore e di sviluppo della manovra finanziaria, non solo, non è stato intaccato, ma appare perfino rafforzato, sia pur lievemente. Infatti, a fronte di una crescita del volume lordo della manovra durante l'esame parlamentare fino all'importo di circa 15 miliardi di euro contro gli 11 iniziali, l'impatto, tanto in termini di saldo netto da finanziare, quanto in termini di indebitamento netto, è perfino migliorato. Il saldo netto da finanziare è infatti migliorato per circa 470 milioni di euro per il 2008, 509 milioni per il 2009, 270 milioni per il 2010. Di analoga entità è il miglioramento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, che - lo voglio ricordare - è il dato rilevante ai fini del Patto di stabilità e crescita e del rispetto dei parametri di Maastricht, il cui importo si è ridotto rispetto al testo presentato dal Governo alle Camere per 380 milioni nel 2008, 583 milioni nel 2009 e 465 per il 2010. Durante l'esame del provvedimento alla Camera è stato trovato il margine finanziario per operare un intervento di restituzione fiscale tra i più sentiti come urgente da una parte, fino ad oggi non sufficientemente considerata, delle famiglie italiane. Nel merito, alle famiglie con almeno quattro figli a carico viene riconosciuta un'ulteriore detrazione ai fini IRPEF pari a 1.200 euro annui, prevedendo anche forme di recupero dell'agevolazione, come nell'ipotesi di incapienza. Sono state stanziate risorse aggiuntive in favore del trasporto pubblico locale, 400 milioni di euro per l'accelerazione degli interventi in materia di viabilità e ferrovie per il finanziamento di nuove misure su trasporti e autotrasporti, per i nuovi interventi in campo sociale e per la gestione delle calamità naturali, oltre a iniziative in materia di sicurezza, ambiente e di investimenti. Con la finanziaria per il prossimo anno si avvia, inoltre, un processo di riforma strutturale del sistema di organizzazione e gestione del trasporto pubblico locale, orientato a riconoscere anche un maggior grado di autonomia finanziaria agli enti territoriali. È in questo senso che va letta l'assegnazione dal 2008 alle Regioni a statuto ordinario di un'ulteriore compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione, i cui importi andranno a finanziare il funzionamento del settore. L'iniziativa è volta a favorire il superamento del tradizionale meccanismo di finanziamento del trasporto pubblico locale, rimesso all'annuale rifinanziamento in sede di finanziaria, promuovendo anche in tale ambito un maggior grado di federalismo fiscale. Nello specifico, viene a tale fine istituito il Fondo per la promozione e il sostegno allo sviluppo del trasporto pubblico locale, le cui risorse sono interamente destinate all'acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale e alla corresponsione di contributi per mutui contratti per lo sviluppo nelle aree urbane degli stessi sistemi di trasporto pubblico. Figura fra questi interventi anche una misura di diretto impatto sulle famiglie, cioè una detrazione *ad hoc* dell'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche per le spese sostenute dai contribuenti per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi del trasporto pubblico locale fino alla concorrenza del suo ammontare nella misura del 19 per cento e per un importo non superiore a 250 euro. Sono state introdotte misure a favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, quale un calcolo più favorevole della pensione diretta spettante alle vittime che abbiano subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa; l'attribuzione di un assegno vitalizio reversibile anche ai figli maggiorenni superstiti, anche se non conviventi; infine, l'esenzione per l'erogazione di medicinali di fascia C agli invalidi vittime di atti di terrorismo e ai loro familiari anche superstiti. Infine - e mi piace ricordarlo - i benefìci in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge n. 206 del 2004, sono stati estesi anche agli eventi terroristici accaduti all'estero a partire dal 1961

anche ulteriori norme in materia di calamità naturali e terremoti; è stato aumentato e definito il contributo concesso ai Comuni delle Marche e dell'Umbria. Vale la pena di menzionare la misura per l'eliminazione del *ticket* sulle prestazioni specialistiche, già introdotta dal Senato su iniziativa parlamentare in prima lettura, con il contestuale reperimento di una copertura finanziaria per oltre 800 milioni di euro, sotto forma di ulteriori tagli di spesa. Una correzione significativa, introdotta da questa Camera, riguarda il previsto limite di 250.000 euro all'utilizzabilità dei crediti d'imposta nello stesso esercizio. A tal A tal proposito, è stata prevista una deroga all'applicazione di tale tetto per le imprese impegnate in processi di ricerca e sviluppo, con un fatturato annuo non superiore a 5 milioni di euro, ubicate nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Molise e Abruzzo. Nel complesso, queste ed altre innovazioni non solo allineano il nostro ordinamento ai sistemi fiscali europei più evoluti, ma spingono le imprese - anche quelle piccole e medie - verso il rafforzamento della capitalizzazione, che a tutt'oggi costituisce un fattore determinante di sviluppo per il nostro sistema economico. La riforma della fiscalità d'impresa delineata dalla finanziaria 2008 avvia il processo di alleggerimento della pressione fiscale sulle imprese, accompagnandolo con una forte semplificazione degli adempimenti contabili e tributari. Non meno rilevanti sono le integrazioni proposte dal Senato alla disciplina per il contenimento dei costi della politica. Rispetto al testo iniziale, che già conteneva importanti misure di riduzione e ottimizzazione dei costi della rappresentanza locale, nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte modifiche orientate, in primo luogo, a contenere le spese per i compensi degli amministratori locali e a ridurre i costi derivanti da duplicazioni di funzioni e dall'utilizzo improprio e disordinato delle forme associative fra enti locali, a partire dalle Autorità di ambito territoriale. Particolarmente incisive sono state anche le norme - introdotte *ex novo* dal Senato - che stabiliscono un tetto di legge alle retribuzioni dei *managers* pubblici, che non potranno superare quella del primo Presidente della Corte di cassazione e si applicheranno a tutti i dipendenti pubblici, sia delle amministrazioni statali sia delle società partecipate e non quotate in Borsa e delle Autorità indipendenti, e la riduzione dei Consigli di amministrazione delle società pubbliche. Un altro importante fronte sul quale si è positivamente speso l'impegno emendativo del Parlamento è relativo alla disciplina del 5 per mille. Una significativa novità, rispetto al testo originario presentato dal Governo, è costituita dalla riproposizione, anche per il 2008, di una disciplina che prevede la destinazione di tale quota del gettito IRPEF a finalità di sostegno ad enti ed organismi che svolgono attività di riconosciuta utilità sociale su indicazione dei contribuenti. A questo proposito, il disegno di legge finanziaria prevedeva originariamente il mero innalzamento del tetto massimo di spesa fissato con riferimento all'ultima disciplina applicabile del 5 per mille. Corrispondendo alle forti aspettative nel frattempo maturate nel Parlamento e nel Paese, il primo ha dunque proposto una nuova disciplina, applicabile alle dichiarazioni dei redditi che saranno presentate dai cittadini nel prossimo anno. Infine, alle politiche per il Mezzogiorno ed alle aree svantaggiate del Paese è dedicato un pacchetto *ad* *hoc* di misure che, in parte, sono del tutto inedite e, per altra parte, ripropongono in forma aggiornata strumenti agevolativi già vigenti. Fra essi, vi è il credito d'imposta per le assunzioni, ripristinato al Senato su iniziativa parlamentare. Nel merito, si prevede che ai datori di lavoro che nel 2008 incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratti a tempo indeterminato, assumendo lavoratori nelle Regioni Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, Basilicata, Abruzzo, Sardegna e Molise, sarà concesso, per il triennio 2008-2010, un credito d'imposta pari a 333 euro al mese per ciascun lavoratore assunto. E per l'assunzione di lavoratrici, il credito d'imposta sale a quota 416 euro al mese. In questo senso, si inseriscono anche le misure mirate a superare il *gap* infrastrutturale che tuttora condiziona lo sviluppo locale. Tra queste, segnalo le disposizioni per l'ammodernamento ed il potenziamento dei collegamenti ferroviari sulla linea Pescara-Roma, tra Avezzano e Roma, con lo stanziamento di 56 milioni di euro all'anno per il triennio 2008-2010, nonché le misure per il potenziamento della metropolitana leggera dell'Aquila, per un importo di 12 milioni di euro per l'anno 2008, e quelle per i Giochi del Mediterraneo. In conclusione, signor Presidente, il disegno di legge finanziaria per il 2008 che ci accingiamo ad approvare in via definitiva - nonostante l'oggettivo appesantimento di nuove norme, subito durante l'esame parlamentare - deve ritenersi un positivo punto di sintesi tra l'originaria proposta del Governo e le istanze emendative emerse in Parlamento. A restare fermo, Presidente, è il comune denominatore costituito dalla triade di sviluppo, risanamento ed equità sociale che connota le politiche economiche e finanziarie di questa legislatura.

Signor Presidente, mi permetta di aprire questa mia brevissima replica aggiungendo, a quella del senatore Bonadonna, la mia espressione di solidarietà nei confronti del ministro Padoa-Schioppa, destinatario, poche ora fa, insieme a due suoi colleghi di Governo, di un anonimo messaggio minatorio. Mi permetta, inoltre, signor Presidente, di ringraziare tutti i colleghi della 5a Commissione e dell'Assemblea per l'attenzione, la fattiva collaborazione ed il confronto propositivo. Dopo tre interventi sul bilancio di previsione dello Stato non ho molto da aggiungere a quanto già detto e registrato. Sui contenuti del disegno di legge n. 1818-B mi limito a sottolineare, ancora una volta, come le modifiche apportate dalla Camera si concretizzino esclusivamente in un miglioramento dei conti pubblici, con una riduzione della spesa complessiva ed un miglioramento di 471 milioni del saldo netto da finanziare. Il giudizio finale sul bilancio, quindi, non può che essere positivo.

informazioni vere, in tempi reali, e della capacità di leggerle, di interpretarle ed elaborarle con spirito critico. Di questo si nutre una democrazia quotidiana e partecipata, una democrazia che non si assoggetti alle dinamiche economiche di un mercato inintelligibile o sfrenato, ma che invece aspiri, nel rispetto della libera volontà di azione dei soggetti economici, a ricondurre verso il bene comune l'azione economica delle istituzioni rappresentative, sia con scelte regolative, sia con scelte operative, investendo risorse, energie ed intelligenze. Coniugare economia e democrazia è un'ambizione alta, una sfida politica lanciata a tutti noi, che mi auguro vorremo raccogliere e provare a vincere.

della quantità di spesa che questo provvedimento comporterebbe, dell'aumento della stessa, dei problemi di copertura, dell'occasione mancata per il risanamento e quant'altro: tutti argomenti che abbiamo ascoltato nel corso

di primo piano, il debito cresceva, la spesa pubblica cresceva, il *deficit* cresceva e l'Unione Europea aveva aperto

ed esatte. Si poteva fare di più? Lo abbiamo detto dall'inizio: certo che si poteva fare di più sul fronte del risanamento, ma il Governo, il Parlamento, la maggioranza hanno deciso di garantire un andamento progressivo del percorso di risanamento, nel rispetto degli impegni internazionali e per fare qualcosa per il Paese, qualcosa di cui il nostro Paese, le nostre imprese, i nostri cittadini avevano bisogno. Era necessario o no fare la riforma della fiscalità d'impresa nel senso che è stato fatto e che conosciamo bene? Era necessario o no fare qualcosa per la casa, finalmente una politica per la casa, con numerosi strumenti che sono stati esattamente allocati dentro la legge finanziaria? Fare qualcosa per i più deboli, finanziare il protocollo sul *welfare*, abolire i *ticket*, rifinanziare l'8 per mille, il 5 per mille, il Fondo per i non autosufficienti? Si doveva dare o no una risposta al precariato, a quel fenomeno che si è rigonfiato nel corso di questi anni, in particolare nella pubblica amministrazione, a causa delle politiche negli ultimi anni? Si doveva dare o no una qualche risposta alle enormi problematiche dell'ambiente, dell'energia, così come abbiamo puntualmente fatto in misura apprezzabile con la legge di cui stiamo discutendo, e dare le tante altre risposte di cui il nostro Paese aveva bisogno? Passiamo all'esplosione della spesa. Ho detto questa mattina e ribadisco (è stato detto autorevolmente dal Governo) l'aumento della manovra lorda non ha comportato mutamento dei saldi, che anzi sono migliorati: perché negate questo? Perché negare che negare che i saldi sono migliorati e che mai come quest'anno il Parlamento si è fatto carico di ricercare coperture attraverso riduzioni di spesa, una diversa allocazione della spesa e, appunto, riduzione della spesa dai 4,7 miliardi iniziali ai 5,7 miliardi al Senato, ai 7,9 miliardi alla Camera, 3,2 miliardi di risparmi in più di quelli ipotizzati all'inizio del percorso della legge finanziaria? Tra questi risparmi spiccano le misure sui costi della politica. Perché si vuole tacere che si è fatto, su questo tema, quello che non si era mai fatto, intervenendo sulle indennità di noi parlamentari, sulla composizione del Governo, sulle consulenze, sui *manager*, sulle comunità montane, sugli enti locali, sugli enti intermedi, sulle società pubbliche, sulla gestione degli immobili pubblici, sui servizi della pubblica amministrazione? È stato stimato un miliardo di risparmio. Quando mai si era fatto tanto, in termini, appunto, di rigore e di adozione di misure che i cittadini si aspettavano?

all'entità, alla qualità, alla consistenza della manovra. Ciò che è certo è che anche con questa manovra proseguiamo con il percorso virtuoso di politica economica e di bilancio di questo Governo e di questa maggioranza. Con tale convincimento profondo credo che possiamo approvare questi strumenti, nella consapevolezza e con la coscienza di aver fatto ciò che si poteva fare nell'interesse del Paese. Vorrei ringraziare tutti per il lavoro che è stato fatto: un lavoro molto intenso

. *Signor Presidente, colleghi,* sentendo gli interventi dei colleghi della maggioranza, che hanno tutti illustrato la bontà dei plurimi contenuti di questa finanziaria, ho avuto come la sensazione di sentire una sorta di catalogo di Leporello, nel quale venivano indicate le conquiste vere o presunte di questa finanziaria, ma credo che, come nell'opera

Signor Presidente, onorevoli senatori, la manovra di finanza pubblica che giunge in seconda lettura nell'Aula del Senato è stata oggetto, in questi mesi, di un ampio dibattito nelle Commissioni e nelle sedute plenarie dei due rami del Parlamento. Anche i mezzi di informazione hanno puntualmente informato il Paese sui contenuti generali della manovra e sui suoi aspetti più significativi. Malgrado la farraginosità del processo, credo si possa affermare che c'è ormai piena consapevolezza delle motivazioni sottostanti alle diverse iniziative contenute nella proposta di bilancio. Una legge così complessa e articolata come la finanziaria, che influisce direttamente sulla vita di milioni di cittadini, non può non essere oggetto di ampio confronto. Quest'anno, pur con i limiti delle attuali procedure che impongono una corsa contro il tempo, la discussione è stata particolarmente ampia e ordinata. Nella mia replica non descriverò nel dettaglio la manovra di bilancio. Mi soffermerò, come di consueto, su alcune delle questioni emerse nel dibattito odierno che ho avuto la possibilità di seguire dagli uffici del Ministero e su alcuni aspetti sollevati in questi giorni in merito alla dimensione finanziaria della manovra. La finanziaria di quest'anno rappresenta un ulteriore passo della strategia di politica economica che il Governo ha messo in atto per sbloccare quell'intreccio perverso tra bassa crescita, ampio disagio sociale e instabilità macroeconomica nel quale l'Italia si trovava all'inizio della legislatura. Dopo lo straordinario sforzo della seconda metà degli anni '90, quando il *deficit* pubblico si ridusse dal 10 per cento del prodotto interno lordo del 1993 allo 0,8 per cento del 2000, vi è stato un nuovo, progressivo deterioramento. Il *deficit* tornò nel 2005 a livelli che non si erano più visti da un decennio. Il prodotto per occupato, che nell'Unione Europea a quindici è - pur modestamente - cresciuto durante la prima metà del decennio, in Italia è addirittura diminuito: la produttività oggi è inferiore a quella registrata nel 2000. Il senso di incertezza che inquieta le giovani generazioni, l'aumento del divario tra lavoratori protetti e non protetti, le persistenti divergenze di condizioni economiche e sociali tra le regioni del Paese rendono davvero sofferte le condizioni di vita di ampie fasce della popolazione. Questa era la situazione all'inizio del 2006. E forse è acconcio ricordare le parole scritte più di sessant'anni fa da lord Baden Powell, il fondatore dello scoutismo. Egli così spronava: «Preoccupatevi di lasciare il mondo un po' migliore di come lo avete trovato». Onorevoli senatori, nessuno può conoscere con certezza gli effetti di un'azione di politica economica, ma non deve mancare la costante volontà di operare per migliorare le condizioni del Paese. Per questo abbiamo inteso farci carico dell'intreccio perverso di cui dicevo, accettando il rischio della impopolarità di alcune scelte. Abbiamo scartato la strada del contrasto con i *partner* europei, della violazione delle regole condivise. Non siamo ricorsi a finanza fantasiosa (64 miliardi di misure temporanee sul bilancio tra il 2002 e il 2005), perché quella è una scelta miope e perdente. Il*deficit* pubblico va ricondotto a livelli permanentemente bassi, in modo da favorire la discesa del rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo. Discesa che non può non essere graduale, se non vogliamo lasciare irrisolti i problemi del basso livello e della qualità del capitale materiale e immateriale e delle inuguaglianze sociali. Questa manovra di bilancio interviene dopo diversi provvedimenti di legge rilevanti per la politica economica: il decreto-legge del giugno 2006, la manovra correttiva dello scorso anno, i decreti di luglio e settembre di quest'anno, tutti indirizzati a perseguire il triplice obiettivo della stabilità macroeconomica, della riduzione dell'ineguaglianza sociale, dell'aumento delle potenzialità di crescita. Le condizioni di finanza pubblica per il 2007 e quelle previste, a legislazione vigente, per il 2008 permettono, senza deviare dal sentiero del risanamento, una riduzione delle entrate per circa 2,4 miliardi di euro e un aumento delle spese di 3,7 miliardi di euro. I principali interventi riguardano, dal lato delle entrate: l'aumento della detrazione ICI, le semplificazioni fiscali, la riduzione delle aliquote marginali IRES e IRAP. Dal lato delle spese: maggiori forze impiegate nella sicurezza dei cittadini, del territorio e dell'ambiente; certezza di risorse stabili per sviluppare il trasporto pubblico locale; norme e mezzi a favore dell'occupazione; azioni volte a ristabilire sobrietà nella politica nazionale e locale. Ecco, in sintesi, gli elementi qualificanti della manovra. È falsa la rappresentazione offerta all'opinione pubblica di una manovra finanziaria stravolta rispetto alla sua impostazione iniziale. Nessuno stravolgimento è avvenuto. Le linee portanti della proposta di settembre sono rimaste intatte. Anzi, escono rafforzate. La dimensione della manovra non è cambiata nei due passaggi parlamentari. L'effetto sul saldo primario è passato da 6 miliardi e 478 milioni di euro del testo licenziato dal Consiglio dei ministri ai 6 miliardi e 503 milioni di euro del testo approvato dal Senato, ai 6 miliardi e 80 milioni di euro del testo approvato dalla Camera dei deputati. Dunque, la manovra oggi in discussione ha ridotto, non aumentato - come si è voluto far credere in questi giorni - il suo impatto sulla finanza pubblica per 400 milioni di euro rispetto alla versione iniziale. In particolare, nei passaggi parlamentari le spese nette sono diminuite - non aumentate - di quasi 200 milioni di euro. Si tratta comunque di variazioni marginali, che confermano l'invarianza dell'impianto. Con questa legge finanziaria rispettiamo gli impegni assunti con Bruxelles e distribuiamo risorse ad ampie fasce di cittadini. Tutto ciò è stato reso possibile non solo dalla straordinaria azione di contrasto all'evasione fiscale e al lavoro nero, ma anche dal controllo stretto della spesa pubblica. Ringrazio il senatore Enriques per aver ricordato come gli andamenti della spesa siano rientrati in una dinamica accettabile. I prossimi mesi ci vedranno impegnati ad impostare la conduzione della finanza pubblica per i prossimi tre anni. È necessario operare da subito affinché ci siano comprensione e condivisione, le più ampie possibili, per realizzare un contenimento della spesa pubblica. Non possiamo ripetere quello che è avvenuto nella scorsa legislatura: un aumento immotivato, strutturale, qualitativamente mediocre, incontrollato della spesa pubblica. Ho ricordato qualche giorno fa alla Camera dei deputati come la spesa primaria corrente sia cresciuta, dal 2001 al 2005, di 120 miliardi di euro, raggiungendo il livello *record* del 40 per cento del prodotto interno lordo. Il treno in corsa è stato frenato nei primi due anni della legislatura; nei prossimi tre anni va arrestato, l'unico modo per dare ai giovani un futuro meno incerto. Andrà profondamente modernizzata la pubblica amministrazione, dovranno essere ridotte le inefficienze negli ospedali, nelle scuole, nei Ministeri, negli uffici delle amministrazioni locali, nei tribunali. Andrà ripensato il pubblico impiego, puntando a uno snellimento delle strutture ridondanti e potenziando quelle più importanti in termini di servizi ai cittadini. Il tempo è maturo per valorizzare i funzionari pubblici che quotidianamente operano in servizi essenziali per la collettività; ma è anche il momento di chiedere una più attiva partecipazione al cambiamento. Vorrei che si uscisse dalla tutela delle rendite di posizione e che uno scatto di orgoglio ci facesse uscire dai cantucci piccoli e meno piccoli nei quali ci si è rifugiati in questi anni. Tutti devono farsi parte attiva della riorganizzazione del pubblico impiego. Il senatore Villone penso sia d'accordo con me che solo attraverso un migliore funzionamento della pubblica amministrazione si possono determinare i giusti aumenti di stipendi e che solo riconoscendo di più il merito si possono moltiplicare le energie dei dei tanti onesti funzionari pubblici. Quanto sto dicendo significa che le risorse non possono, non devono essere reperite attraverso tagli che non differenzino tra realtà molto diverse una dall'altra. Si spendono ogni anno circa 350 miliardi di euro per scuola e università, sanità, pubblico impiego, trasferimenti alle imprese, difesa, ordine pubblico. Per un ammontare di risorse così cospicuo mancano un'analisi e una valutazione approfondita, pur se sono presenti singole indagini nell'ambito delle amministrazioni: non sono infrequenti i rapporti inviati al Parlamento, redatti sulla base di disposizioni di legge, al fine di monitorare specifiche componenti di spesa pubblica. Di fatto, tali indagini rimangono nell'ambito di circuiti molto ristretti e non hanno ricadute sull'allocazione delle risorse finanziarie. Purtroppo l'analisi della spesa pubblica in Italia è in netto ritardo rispetto ad altri Paesi europei che usano da tempo metodologie avanzate di pianificazione e valutazione. Migliorare l'efficienza e la qualità del denaro pubblico erogato è diventato un imperativo non più procrastinabile. Lo si può obbedire solo intervenendo sui meccanismi profondi di generazione della spesa, rivedendo le priorità in ciascun settore, per il recupero di risorse da reinvestire in spesa migliore e in riduzione del debito. Dovrà poi continuare con maggiore vigore la restituzione fiscale cominciata quest'anno. Tale azione sarà tanto più incisiva quanto più diventerà strutturale il recupero di gettito. I dati sul 2007 sono confortanti e confermano il cambiamento di tendenza cominciato nel 2006. Secondo le ultime valutazioni, pervenute ieri mattina anche all'Aula del Senato, le principali imposte mostrano un andamento più che positivo a conferma del recupero di base imponibile. Tali dati, coerenti con le previsioni formulate nella Relazione previsionale e programmatica, ci fanno essere moderatamente ottimisti sul fatto che l'anno in corso chiuderà con un rapporto tra deficit e PIL inferiore al 2,4 per cento stimato a fine settembre. Sarà comunque necessaria ancora un'azione vigorosa per rendere tali andamenti strutturali nel tempo. Con il volume ancora ampio di economia sommersa c'è spazio per una riduzione delle aliquote fiscali che non impedisca un aumento di gettito e che non penalizzi i conti pubblici. Vengo ora ad alcune considerazioni più puntuali sorte nel corso del dibattito. La senatrice De Petris, il senatore Albonetti e il senatore Vegas ci ricordano come la finanziaria contenga misure a volte stravaganti e come sia necessario riformare la sessione di bilancio. Benissimo: spero che durante il 2008 si riesca a intervenire con atti condivisi da maggioranza e opposizione su procedure e regolamenti in modo da rendere più fluido il processo e limitare la finanziaria a poche ed essenziali misure. L'azione in questo senso spetta al Parlamento, non al Governo. Il senatore Tecce ha sottolineato un aspetto piccolo, ma non marginale, contenuto nella finanziaria: la possibilità di anticipare agli enti locali le risorse stanziate con la finanziaria per attivare politiche sociali senza aspettare il lungo *iter* che spesso porta i Comuni a disporre solo verso la fine dell'anno dei mezzi per attivare essenziali servizi per le fasce più povere. Questo permetterà una migliore programmazione delle attività migliorando, spero, il tipo di servizio offerto. Mi auguro che, attraverso vie amministrative, si lavori nei prossimi mesi per rendere più fluidi i flussi di risorse verso gli utenti finali in modo da rispettare pienamente le deliberazioni del Parlamento. Il senatore Asciutti sostiene che al Governo non interessa il risanamento del Paese. Credo abbia sbagliato interlocutore. Gli suggerisco di informarsi meglio presso chi ha fatto sì che il debito pubblico in rapporto al PIL sia ripreso a crescere nel 2005 dopo un decennio di costante discesa, che il *deficit* sia salito oltre il 4 per cento, che la spesa pubblica sia cresciuta senza freni. La senatrice Bonfrisco, con molta enfasi, fa un "attacco" alle tasse. Le chiedo quale alchimie finanziarie abbia in mente per mantenere in servizio i poliziotti, i vigili del fuoco, gli insegnanti, per illuminare le strade. E poi la senatrice dovrebbe chiedersi perché le tasse sono dovute aumentare. Le offro una risposta: sono salite perché erano dissennatamente scese per alcune categorie di cittadini negli anni precedenti, senza una strategia di contenimento della spesa che permettesse di snellire l'apparato pubblico. Il senatore Izzo indica come un miglioramento l'emendamento da lui proposto, e inopinatamente approvato qui in Senato, che rinviava al 2010 l'attuazione della riforma del Ministero dell'economia e delle finanze, limitandola alle Province con popolazione superiore ai 250.000 abitanti. Non vedo francamente quale fosse il miglioramento: si rinviava la riforma e se ne riduceva la portata. Il mondo, senatore Izzo, è cambiato rispetto a quando vennero istituiti quegli uffici e ciò richiede, anzi impone, una riorganizzazione. Chiuderanno 80 uffici su 206; non mi sembra di aver svuotato il territorio della presenza del Ministero. E poi mi permetto di ricordare ai senatori che lo stesso personale - peraltro qualificato - potrà essere più utilmente coinvolto all'interno degli stessi territori in servizi che hanno diretta utilità per le comunità locali. Signor Presidente, onorevoli senatori, a chi gli chiedeva se valesse la pena di rischiare per una causa giusta, Kant rispondeva: «Coloro che dicono che il mondo andrà sempre così come è andato finora contribuiscono a far sì che l'oggetto della loro predizione si avveri». Riportai questa frase nel DPEF del luglio 2006. La manovra di bilancio rappresenta un tassello di un complicato mosaico di azioni legislative, amministrative e di cambiamenti culturali necessari per modificare la direzione di marcia del Paese. Sottolineo: un tassello. Non si deve, non si può imputare alla manovra di bilancio tutta la responsabilità o tutto il merito di un eventuale successo o insuccesso dell'azione di politica economica del Governo. Il mosaico sarà completato quando l'Italia tornerà a crescere in maniera sostenuta e duratura. Il risanamento dei conti pubblici e il miglioramento della qualità della spesa sono condizioni essenziali. Un bilancio prossimo al pareggio permette una rapida riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo e dunque un risparmio, per minor spesa per interessi sul debito pubblico, che può essere destinato alla riduzione delle tasse o a spesa produttiva. Inoltre, favorisce la creazione di un miglior clima di fiducia fra gli operatori economici, con effetti benefici sui consumi e gli investimenti. Il settore pubblico in Italia è ampio, molto ampio. Un miglioramento della sua produttività è indispensabile perché si innalzi la produttività complessiva del Paese. Spesa pubblica di qualità, per una economia più competitiva. Spesa pubblica contenuta, per liberare risorse. Questa è la strada per ridare slancio all'economia italiana.

che con l'approvazione dei singoli articoli si intendono approvati anche le tabelle, i quadri generali, gli allegati e gli elenchi richiamati dagli articoli stessi e riportati nello stampato 1818-B (con la Terza Nota di variazioni). Passiamo quindi all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. Passiamo alla votazione

Passiamo alla votazione dell'articolo 5, con l'annessa tabella.

su uno degli articoli del bilancio, dal porre una domanda, che rivolgo alla Presidenza, perché così deve essere, ma chiedo ma chiedo che la Presidenza la rivolga al Ministro dell'economia. Visti tutti gli insulti che ha rivolto al generale Speciale, signor ministro Padoa-Schioppa, che ha avuto la dignità di dimettersi...

ultimare gli interventi dei parlamentari. La mia domanda era molto semplice. Mi perdoni, Presidente, ma la domanda che volevo rivolgerle e che l'Aula vuole rivolgere al Ministro, viste le cose che abbiamo detto è la seguente: quando ci pregia delle sue dimissioni, signor Ministro? Grazie.

è assolutamente irrituale che il Presidente intervenga durante una dichiarazione di voto ed interrompa un senatore che, nell'ambito regolamentare, dice ciò che crede

a voi! Credo che i princìpi fondamentali della democrazia dovrebbero essere difesi da tutti. Basta che uscite dall'Aula e capite l'aria che tira nel Paese; non credo che la prossima volta sarete voi in maggioranza. Quindi, quello che sto dicendo probabilmente serve più a voi che a noi. Presidente - glielo dico con la maggior pacatezza possibile - la prego di non interrompere i miei colleghi quando intervengono in un ambito perfettamente regolamentare, anche perché, se magari riusciamo ad innervosire il Ministro, ci gratificherà dei suoi sorrisi, che ormai sono diventati famosi in quest'Aula.

nei mesi scorsi sul più alto esponente della Guardia di finanza, rassegni qui, oggi, irrevocabili dimissioni e non che noi aspettiamo e speriamo che le dia. Pensiamo che ciò sia indispensabile per avere un briciolo di dignità sia come Governo

ha evidenziato i risultati ottenuti - ha dichiarato - nella lotta all'evasione. Poiché il generale Speciale, comandante della Guardia di finanza, ...Voi prendete l'elicottero anche per andare ad Ischia ed il signor vice ministro Visco si fa accompagnare da una motovedetta della Guardia di finanza nei siti archeologici. Quindi, tacete e non parlate. Lasciamo perdere!

i risultati ottenuti dal generale Speciale in tale ambito. Allora, signor Ministro, il generale Speciale era un generale fellone, che stava dalla parte degli evasori, o era un generale che svolgeva il suo lavoro positivamente e con grande professionalità? e con grande professionalità? I risultati ottenuti infatti contrastano con le parole pronunciate in Aula da un Ministro abituato a mentire su questa e su altre situazioni.

Qui abbiamo sentito di tutto, da quelli che fanno l'apologia e il panegirico della Rivoluzione di ottobre a quelli che fanno lo stesso su altri argomenti e nessuno è mai intervenuto

Abbiamo qui un Ministro, professore universitario, che ci ha descritto un personaggio come assoluto delinquente, anche se il giorno prima voleva destinarlo alla Corte dei conti; che è venuto in Commissione vigilanza RAI a dire che quell'altro era un totale incapace, che non rispondeva

Spagna, della Grecia e del Portogallo era come parlare dell'Africa dal punto di vista economico, non certo per il rispetto delle persone, ci mancherebbe sia per loro, che per gli africani. Oggi scopriamo che ci stanno superando mentre tale evento

ad un distretto tedesco e alla regione di Parigi, ha il più alto PIL *pro capite* del mondo; e adesso ci troviamo attaccati ad un carrozzone statale che ci fa finire dietro la Spagna.

in occasione del dibattito che si svolgerà in quest'Aula nel mese di gennaio, dove ci auguriamo di ascoltare le parole del Ministro o del Presidente del Consiglio, come è di rito, per esporre le motivazioni del Governo che inviteranno la maggioranza

quella data in cui cercheremo di far chiarezza. Inoltre, ci attendiamo anche da lei, signor Ministro, una chiarezza che, punto per punto, le possa consentire di difendersi dalle motivazioni dei giudici amministrativi e non del presidente Schifani, né di altri.

giuridiche che attengono alla gestione del procedimento di revoca da funzioni pubbliche. Inoltre, un'altra contraddittorietà è averlo proposto per la Corte dei conti; non staremo, però, a parlare della sentenza e mi auguro che a quella data ella abbia letto e studiato attentamente le motivazioni della sentenza. quello che lamento, signor Presidente, è un altro dato. Siamo preoccupati perché in quest'Aula si verificano fatti emblematici per la vita del nostro Paese.

Apprendiamo, in data odierna, che il Governo ha deciso di far decadere l'intero provvedimento che atteneva alla sicurezza dei cittadini perché si è reso conto di quell'errore, ma anche perché si è reso conto che probabilmente avrebbe trovato forte difficoltà nella promulgazione di quel decreto contenente errori. Pertanto, anziché modificare, ablare, togliere, emendare quella disposizione e rimandarla in Senato, che avrebbe avuto tutto il tempo per approvare il decreto senza quella norma,

che non ha tenuto conto dell'appello del presidente Pera che invitava l'Assemblea a tener conto del fatto che la norma conteneva riferimenti errati. Ma vi è di più, signor Presidente; comincio a dirlo sin d'ora, lo farò nei giorni seguenti e faremo anche appelli a cariche autorevoli del nostro Paese. Tra qualche giorno si consumerà un altro strappo, colleghi senatori; come è stato anticipato già ieri in Conferenza dei Capigruppo, saremo chiamati ad un voto di fiducia su un provvedimento che non è la finanziaria, sulla quale quantomeno, in prima lettura, ci siamo confrontati e abbiamo votato in Commissione e in Aula; no, saremo chiamati ad un voto di fiducia sul disegno di legge sul *welfare* e sulla riforma delle pensioni

tanto è vero che il testo arriverà in Aula senza relatore proprio per l'ostruzionismo della maggioranza. Sappiamo il motivo di tutto questo: la maggioranza si sarebbe divisa sui primi emendamenti e si sarebbe ripetuto lo scenario della Camera. arriverà in Aula, signor Presidente, senza che nessun senatore abbia potuto esercitare una funzione di voto in Commissione, e nemmeno in Aula potrà esercitare analoga funzione, se non per passare da quello scranno e dire sì o no al Governo. Signor Presidente, questo è un commissariamento totale e senza precedenti del Senato*. (Applausi dal Gruppo FI).* È un fatto grave, gravissimo, senza precedenti, colleghi dell'attuale maggioranza. E lo dico a voi perché, nella logica di un sistema bipolare, quello che accadrà fra qualche giorno vi dovrebbe preoccupare. Siamo eletti per esercitare le nostre funzioni: una legge importante e strutturale come la riforma delle pensioni postulava e pretendeva necessariamente l'esercizio dell'attività dei parlamentari qual è quella del voto o in Commissione o in Aula, e in prima lettura in particolar modo. A cosa saremo chiamati? A non esercitare la nostra funzione su quel testo: mi dica lei, signor Presidente, se questo è il Senato; se a questo si è ridotto il Senato. Chiedo a lei un gesto di tutela delle nostre funzioni: ora lo chiediamo a lei, domani lo chiederemo al Capo dello Stato.

ministro Visco, stiamo aspettando che entri in vigore questa finanziaria, perché non vediamo l'ora di pagare il nostro contributo, quei pochi centesimi che ci chiedete sul consumo di ogni litro di benzina: non

vorrei ringraziare il Ministro dell'economia per essere presente in Aula, anche perché pare che abbia una particolare dimestichezza con le questioni economiche e numeriche oggetto di questo provvedimento, anche se questa dimestichezza non pare essere condivisa dai colleghi Vegas, Sacconi e Ferrara, che

sia pur rimandando l'appuntamento della chiarezza alla data in cui si discuterà della mozione di sfiducia. Signor Ministro, due giorni dopo il suo intervento sul generale Speciale da molti di noi fu presentato garbatamente, cortesemente e, se si vuole, anche pacatamente un atto di sindacato ispettivo,

nel provvedimento concernente la destituzione del generale Speciale, né tantomeno era ricordato nell'intervento del ministro Padoa-Schioppa.

L'esame degli articoli del disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è pertanto concluso. Onorevoli colleghi, secondo le cadenze stabilite dal Regolamento, la votazione finale del disegno di legge di bilancio sarà effettuata solo dopo la votazione del disegno di legge finanziaria nel suo complesso.

a nome del Governo, autorizzato a ciò dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sulla distinta approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, degli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge n. 1817-B (legge finanziaria 2008), nel testo approvato dalla Camera dei deputati ed esaminato dalla Commissione bilancio del Senato.

una nuova finestra"). Comunico le decisioni della Conferenza dei Capigruppo circa l'organizzazione del dibattito sulle tre questioni di fiducia poste dal Governo sul disegno di legge finanziaria. Avrà iniziò ora la discussione generale congiunta che proseguirà fino alle ore 22. La discussione riprenderà domani mattina dalle ore 9,30 alle ore 10,30 e, quindi, dalle ore 12,30 alle ore 13,30. Resta confermato che la seduta sarà sospesa dalle ore 10,30 alle ore 12,30 in concomitanza con la cerimonia di auguri al Capo dello Stato al Quirinale. generale sulla fiducia, sarà posto all'ordine del giorno il documento della Giunta concernente i reati ministeriali sul quale, dopo la relazione del senatore Manzione, si svolgerà una discussione limitata con un intervento per Gruppo, per non più di 10 minuti, fino alla conclusione del dibattito e quindi eventualmente anche oltre le ore 14. Le votazioni avranno luogo in un secondo momento, come precisato oltre. Nel pomeriggio di domani, giovedì, dalle ore 16 riprenderà, ove non conclusa, la discussione generale sulla fiducia, per la quale sono state ripartite complessivamente quattro ore. Inizieranno poi le dichiarazioni di voto congiunte sulle tre questioni di fiducia e sui voti finali dei disegni di legge finanziaria e di bilancio. La prima chiama avrà inizio non prima delle ore per consentire ai senatori che lo desiderano di recarsi al concerto di Natale previsto dalle ore 17 alle ore 18 presso la Sala della Lupa alla Camera dei deputati. Intorno alle ore 19,30 avverrà la seconda chiama. Sarà quindi tolta la seduta. La terza chiama e il relativo scrutinio avranno luogo venerdì 21 dicembre alle ore 9,30. Subito dopo saranno effettuate le votazioni finali con scrutinio elettronico sul disegno di legge finanziaria e sul disegno di legge di bilancio. Si passerà quindi alla serie di votazioni elettroniche sul documento della Giunta concernente i reati ministeriali, per la cui approvazione è necessaria la maggioranza assoluta. In ogni caso, i senatori che non abbiano partecipato ai voti elettronici potranno comunicare i propri voti in modo palese ai senatori segretari che ne terranno nota in appositi verbali fino alle ore 19. Successivamente riprenderà la discussione generale sul disegno di legge collegato recante il Protocollo sul lavoro e previdenza, con l'intervento del senatore Treu e quindi la replica del Governo. **Calendario dei lavori

Presidente, colleghi, la finanziaria sulla quale il Governo ha posto la fiducia perché sia licenziata definitivamente in tempo utile dà il segno della direzione che da gennaio il centro-sinistra può e deve prendere con maggiore determinazione. Abbiamo trovato nell'intenso lavoro del Governo, del Senato in prima lettura e infine della Camera, quel segno di una inversione di tendenza che consentirà di avviare una vera redistribuzione della ricchezza nel nostro Paese a favore delle fasce più deboli e dei lavoratori. Cominciamo ad affrontare una vera e propria emergenza, la perdita del potere di acquisto dei cittadini sia sul versante dei salari che dei prezzi, come ricordatoci addirittura dal Governatore della Banca d'Italia. La decisione di rendere ancora più cogente ed immediatamente operativa la riduzione del carico fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, attraverso le risorse recuperate dalla lotta all'evasione fiscale, è una scelta positiva che risponde ad una determinata politica. La lotta all'evasione è una necessità nazionale che fa vivere meglio tutti i cittadini a partire dai più deboli. Rafforzare l'unità di questi due interventi, un aumento del salario tramite la riduzione delle tasse e l'impegno serrato perché tutti paghino le imposte dovute, è un segno di coerenza politica. Ma, come noto, il potere d'acquisto non ha solo la variabile di quanto ciascuno percepisce: il lato delle entrate. Ci sono anche le uscite, cioè quanto ciascuno spende per i beni primari. Anche qui rileviamo scelte importanti contenute nella legge finanziaria: la sterilizzazione delle accise sui carburanti, una più valida norma di estinzione dei mutui, l'introduzione del Garante dei prezzi, che integra quell'osservatorio per il comparto agroalimentare che è stato introdotto dal Senato in prima lettura, sono tutte misure che puntano ad abbattere il costo della vita. Dopo una lunga fase di aumenti pesantissimi non registrati dalle statistiche dell'inflazione ma percepiti come evidenti dalla larga parte dell'opinione pubblica, oggi segniamo un'inversione di tendenza beneaugurate. La perdita di potere d'acquisto è ancora più visibile sulla casa, anche in ragione dell'impazzimento dei mutui a tasso variabile. Su questo sensibile terreno la Finanziaria interviene con il fondo di solidarietà per i mutui prima casa. Più soldi alle famiglie e ai lavoratori, un fisco equo e rigoroso e una politica più sobria. La scelta di mantenere sostanzialmente immutate le norme che noi abbiamo introdotto in prima lettura sui costi della politica e in particolare quella sui *manager* pubblici, ad eccezione di Banca d'Italia, Autorità e RAI, conferma una linea di sobrietà che è riuscita a resistere a forti pressioni contrarie che si sono evidenziate nelle scorse settimane. Vorremmo poi, in questa disamina degli aspetti qualificanti della manovra, richiamare l'attenzione sulla riforma delle modalità di gestione per i beni confiscati alle mafie. Questa misura, insieme all'equiparazione delle vittime di mafia alle vittime di terrorismo, consente di affrontare con maggiore efficacia e celerità l'uso dei beni. E' un messaggio che non vogliamo passi sotto silenzio. Ogni volta che un bene confiscato resta, magari per anni, abbandonato, che si tratti di un terreno agricolo o di un'impresa, si produce uno scoramento nei cittadini onesti. Per dare una risposta positiva a tutti questi, oggi mettiamo in moto i primi strumenti: i beni confiscati alle mafie devono diventare subito un patrimonio riconsegnato alla collettività. La lotta alla criminalità organizzata, come spesso abbiamo verificato in Commissione Antimafia, è sicuramente fatta dal lavoro quotidiano e coraggioso delle Forze dell'ordine e della magistratura, a cui va tutta la nostra stima e solidarietà, ma è fatta anche da tanti interventi di prevenzione e cultura della legalità, dalle scuole all'uso sociale dei beni confiscati. E anche su questo terreno non abbiamo intenzione, e nessuno deve avere intenzione, di abbassare la guardia. Se questi sono alcuni aspetti positivi tra i contenuti della Finanziaria, mi sembra opportuno far cenno anche ad altri meno postivi, che richiederanno approfondimenti e successivi interventi correttivi, resi ora impossibili da scadenze ordinamentali. Prendiamo atto di come sul terreno dell'università e della ricerca neppure la Camera sia riuscita a migliorare la pur valida proposta trasmessa dal Consiglio dei ministri al Parlamento. Mentre per la scuola si è scelto, giustamente, di assicurare le risorse per i rinnovi contrattuali, e la Camera ha confermato, facendolo proprio, lo stanziamento di 40 milioni di euro per aumentare le borse dei dottorandi, per l'università assistiamo ad una riduzione di circa 90 milioni di euro dell'aumento previsto del fondo ordinario. Ancor più grave è stata poi la scelta di escludere dalla stabilizzazione prevista dal Senato il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento e di ricerca nelle università e negli enti. Quella decisione di un percorso efficace di stabilizzazione è una scelta che noi rivendichiamo, e il punto semmai sarà quello di passare da un intervento che si limita al settore pubblico ad un'azione incisiva e generalizzata che cancelli la precarietà dall'orizzonte di vita delle giovani generazioni. Ma proprio perché rivendichiamo quella scelta del Senato, critichiamo nel merito e nella forma l'esclusione di cui sono oggetto i ricercatori e i professori universitari a contratto. Nella forma perché si affiancano queste figure agli uffici di diretta collaborazione della politica, che godono di un rapporto fiduciario, mentre professori e ricercatori hanno tutt'altro tipo di rapporto e selezione. E nel merito perché è inutile continuare a sostenere ad ogni convegno la centralità della ricerca e della formazione universitaria, quando affidiamo queste funzioni fondamentali per lo sviluppo del Paese a contrattisti precari pagati poche centinaia di euro al mese. Abbiamo trasformato la figura del docente universitario in una sorta di secondo lavoro per soggetti che vivono di altro e a titolo poco più che volontario formano la futura classe dirigente. Addirittura ci sono casi di professori a contratto che assommano quattro o cinque corsi in università di Regioni diverse, con più tempo passato in treno che nelle aule universitarie. Non cogliere che nella stabilizzazione di questi soggetti stava una leva fondamentale per la qualificazione del sistema universitario, prima ancora che la garanzia di diritti basilari, è segno di una miopia alla quale spero che, in un futuro provvedimento, potremo porre rimedio. Questi elementi che dovranno essere corretti non inficiano il nostro giudizio generale: con questa finanziaria si avvia un nuovo inizio, al quale il Governo dovrà dare continuità, per assicurare più diritti e più salario a chi lavora e per ridurre il costo della vita per tutti i cittadini. E, di fronte a questi risultati che avranno effetti concreti ed immediati, il ricorso alla fiducia è un costo meno pesante delle tante fiducie alle quali abbiamo assistito nella scorsa legislatura.

Replico in maniera puntuale, spero anche garbata, ma ferma, alle dichiarazioni del ministro Padoa-Schioppa. Mi dispiace di dover iniziare con una nota di rammarico

È presente quando si tratta di votare, cioè in un momento in cui, francamente, anche se non ci fosse nessuno ne avvertirebbe la mancanza; sostiene che ha seguito nel pomeriggio dal Ministero Ministero una certa parte del dibattito che è avvenuto in Aula. Non sono certo all'altezza di dare consigli ad un Ministro, figuriamoci, ma gli consiglierei, come sta facendo il sottosegretario Sartor lodevolmente - immagino con una delega esplicita del Ministro esplicita del Ministro - di venire qui ad ascoltare anche i senatori di fila, come sono io, e non solo i Capigruppo, gli ex Ministri, coloro che fanno notizia, che vanno sulle agenzie e disturbano i titoli dei giornali. magari proprio da chi è nuovo in quest'Aula può venire finalmente una parola diversa, forse più persuasiva e credo anche più trasparente e serena

perché da un dialogo più franco e diretto, guardandoci negli occhi, credo che potrebbe guadagnare esperienza e magari anche un pizzico di simpatia che gli eviterebbe certi

Mi rivolgo a lei, signor Sottosegretario, non considerandola certamente un gregario di secondo piano. Lei ha seguito tutto il dibattito e sicuramente è più competente e a conoscenza delle nostre problematiche del Ministro, che è preso da molte altre questioni "speciali", mettendo tra virgolette, con un pizzico di ironia, questo che non è un aggettivo. Il Ministro ha sostenuto che intende spezzare lo sbilancio tra la bassa crescita e il ridotto sviluppo sociale; come può farlo se pochi istanti dopo ha annunciato la diminuzione costante e irrefrenabile del prodotto interno lordo? Ciò è dimostrato, come molti hanno ricordato durante il dibattito, dal sorpasso, che ci fa arrossire, della Spagna nei nostri confronti. sarebbe meno sorprendente per molti se avessero seguito il percorso virtuoso che la Spagna ha compiuto negli ultimi 10-15 anni, ad esempio per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi strutturali europei e dei 1.000 programmi che l'Unione Europea mette a disposizione dei Paesi più più svegli, attenti e pronti a recepirli. Se girate la Spagna, o se lo aveste fatto da 15 anni a questa parte, avreste notato su ogni cantiere spagnolo una bandierina con le dodici stelle dell'Unione

il sorpasso della Spagna non mi ha sorpreso più di tanto, anche se mi abbatte; temo il sorpasso della Grecia che non ha avuto e non ha il *curriculum* della Spagna; inoltre, già sappiamo che sono in corsia di sorpasso, con le freccia già accese e lampeggianti, il Portogallo e la Slovenia e ci va bene che non siano ancora entrate nell'Unione Europea la Croazia e la Turchia. Come si fa a rimediare a questo declino che anche lo stesso Ministro ha definito inarrestabile? Sicuramente tutti dobbiamo rimboccarci le maniche.

ma sicuramente è nebulosa e mette tanta carne al fuoco senza curarsi del fatto che nessuno ha il carbone per accenderlo; senza preoccuparsi delle famose coperture, come direbbero gli esperti di bilancio, quindi molte iniziative annunciate rimarranno incompiute perché non hanno la materia prima, cioè le risorse. Il Ministro ha anche detto che vuole unire alla riduzione delle entrate, con la diminuzione dell'ICI che interessa una minima parte dei cittadini italiani, un aumento delle delle spese. Potrebbe apparire un controsenso, in effetti se non è un controsenso è una sicura contraddizione nei termini. Intanto, al Governo è sfuggito totalmente il controllo dei mercati internazionali, ma anche di quelli nazionali. È sotto gli occhi di tutti la polemica sui prezzi, lievitati oltre ogni ragionevole giustificazione in questi giorni, dopo lo sciopero: è dunque bastato uno sciopero degli autotrasporti per far salire alle stelle i prezzi di moltissimi prodotti sui mercati. Qui manca un controllo del Governo: vi è una responsabilità di chi dovrebbe allertare questi controlli. Ma le contraddizioni, per quanto concerne gli aumenti delle spese, riguardano l'annunciato aumento per la sicurezza: proprio in questo momento, il Presidente della Repubblica respinge - e con veemenza, direi, con un gesto teatrale - il pacchetto sicurezza, bocciando un progetto ambizioso del Governo. Così, ha messo in difficoltà il Ministro competente, Amato, il quale aveva addirittura preannunciato le proprie dimissioni in caso di fallimento di questo pacchetto, che quindi è stato bocciato. Dove e a chi andranno, allora, le risorse annunciate dal Ministro? Ha detto ancora che vuole aumentare la spesa per il trasporto pubblico: ci vuole davvero una bella fantasia, nel momento in cui vediamo le Ferrovie dello Stato in preda ad un dissesto inarrestabile ed assistiamo all'operetta buffa dell'aggiudicazione delle azioni di Alitalia e dell'operazione di soccorso internazionale verso Alitalia. Ci vuole sobrietà, ha detto il Ministro, nella politica locale e statale, ribadendo che anche alle assunzioni di nuovi dipendenti si deve procedere con misura. Oggi troneggia su tutti i giornali l'annuncio che, tra quelle già fatte e quelle che verranno effettuate tra pochi giorni, ammontano a 100.000 le nuove assunzioni nel servizio pubblico. E tutto questo, senza rispondere fino in fondo alle esigenze dei giovani e dei precari e senza avere una prospettiva chiara, al di là di quei giovani e di quei precari delle Regioni messi a posto, ma a scapito di molti altri, che avevano fatto regolare concorso e lamentano ora di essere stati messi in coda. detto ancora il Ministro, poco fa, che il recupero dell'economia sommersa è uno strumento per ridurre la pressione fiscale in futuro: lo sentiamo dire dal primo giorno, dalla presentazione del programma di questo Governo. Capisco che i tempi siano lunghi e sia un'operazione difficile, ma qualcosa sarà pure stato fatto sotto questo aspetto, per questo problema. Perché, allora, non dirci qualche cifra o darci l'annuncio di quanto è stato fatto, senza continuare a dire che il sommerso aiuterà una ipotetica, futura riduzione della pressione fiscale? Ho poi apprezzato anche un certo percorso, uno *slalom* che il Ministro ha fatto tra i vari interventi di centro-destra e di centro‑sinistra, sottolineando alcune affermazioni rilasciate da colleghi

evidentemente, non ho detto nulla di interessante per il signor Ministro. So perché: ho parlato soprattutto, ancora una volta, della montagna. Signor sottosegretario Sartor, mi rivolgo a lei, che porta un nome veneto: ma possibile che la montagna non incontri alcuna considerazione e attenzione da parte di questo Governo? La signora ministro Lanzillotta, che ha la delega in materia, non ha fatto una sola azione a favore delle problematiche di montagna. Da un lato, meno male, signor Sottosegretario: le poche volte che se n'è occupata, come la settimana scorsa, per organizzare la Giornata internazionale della montagna, ha fatto solo disastri. Va detto, inoltre, che il ministro Padoa-Schioppa, ignorando totalmente la mia denuncia ed il mio grido di allarme ed il grido di soccorso da parte delle popolazioni di montagna, ha confermato che, a questo Governo, delle problematiche delle persone che ci vivono non importa nulla. E non sono poche, rappresentano pochi voti. Allora, con un pizzico di malizia (che il nostro collega giustifica sempre come ultima ragione di ogni azione politica), debbo capire che non interessano i voti della gente che vive in montagna; eppure,

ma il Governo continua a non interessarsi della montagna. attraverso lo scellerato emendamento che voleva la soppressione delle comunità montane. Con un solo colpo di accetta violento, più di quello del boscaiolo cha abbatte un abete secolare, la signora Ministro tentava di ridurre a zero le comunità montane, per sostituirle con non si sa bene cosa, pare con delle agenzie collocate a Roma, destinate a raccogliere l'impegno amministrativo e politico di questi Comuni e delle comunità stesse. Non è riuscito il colpo perché alla Camera dei deputati, forse dopo il dibattito che vi è stato in quest'Aula, con evidenti imbarazzi da parte del Governo, si è corretto l'errore. È stata ora assegnata alle Regioni una delega precisa ed esplicita per cui, entro sei mesi, dovranno provvedere al riordino delle comunità montane inserendo, accanto ad indicatori esclusivamente altimetrici, anche indicatori demografici e socio-economici per definire la montanità o meno

Ecco dove il Governo non ha una lucidità di pensiero e non ha mai manifestato una volontà di intervento. È allora davvero un anacronismo che non ci sia il rispetto per la montagna, dove esistono storicamente da sempre istituzioni capaci,

ad una tradizione di impegno civile, politico e amministrativo, un colpo di spugna con un intervento arbitrario che il presidente dell'UNCEM, in un coraggioso articolo apparso oggi su un quotidiano romano ha definito addirittura «un tentativo «un tentativo di colonialismo amministrativo». Certo «colonialismo» è una parola forte, ma in effetti, se fosse riuscita l'operazione che la signora ministro Lanzillotta aveva Lanzillotta aveva tentato di fare, i montanari sarebbero stati considerati come gli abitanti di una riserva indiana, quasi di un ghetto isolato, gente incapace non tanto di intendere e di volere, ma di pensare a se stessa e quindi sottoposti ad una sorta di tutela da parte del Governo centrale. Nel momento in cui il processo del federalismo sotto molti aspetti sta avanzando e sta convincendo anche i più scettici, nel momento in cui le autonomie locali stanno manifestando la bontà della formula, se affidate a persone coscienti, questo Governo centralistico, ancora una volta, propone di cancellare un'esperienza di amministrazione territoriale e di autoresponsabilizzazione della gente per sostituirla con una atto di imperio. Signor Sottosegretario, la prego, porti alla signora ministro Lanzillotta tutto il peso di questa mia forte critica che non cesserò mai di fare e dica al Presidente del Consiglio, che si qualifica mezzo montanaro, di pensare

a osare un po' di più; e, al di là delle contingenze dei singoli articoli e anche delle insufficienze che naturalmente ci sono nella complessiva manovra di bilancio, ci ha esortato a prendere atto che negli anni che ci stanno alle spalle si era registrato un aumento, che lui ha definito incontrollato, strutturale, qualitativamente mediocre della spesa pubblica e a ragionare insieme su come un rigoroso controllo, un migliore utilizzo della spesa pubblica potesse costituire in sé un atto di orgoglio, di riscatto per la valorizzazione dei funzionari pubblici più capaci, dei talenti migliori, per far sì che quei 350 miliardi di euro (mi sembra che abbia così quantificato le grandi dotazioni di spesa: la sanità, l'assistenza, la scuola, la giustizia, l'ordine pubblico e così via), che non sono aumentabili e non saranno significativamente aumentabili nei prossimi anni, possano sì, attraverso la cosiddetta *spending review*, essere fattori di migliore razionalizzazione interna, di crescita, di sviluppo. E come non andare, sentendo le parole del ministro Padoa-Schioppa, al Libro verde sulla spesa pubblica, che è stato importante fonte ispiratrice per il Governo, laddove appunto sosteneva che la difficile sfida del Paese consiste nel combinare l'aumento del contributo del bilancio alla crescita, la progressiva riduzione del carico fiscale sui contribuenti che hanno fatto il loro dovere, l'alleggerimento del debito pubblico. Forse non tutta la struttura del Governo, non tutti i Ministeri, non tutta la maggioranza, insomma forse non è ancora matura la capacità di leggere nella spesa, di redistribuire la spesa e di far sì che questa (che nei grandi comparti è analoga a quella europea, ma non ha la produttività dei fattori di quella europea) venga, per così dire, aggredita nel suo funzionamento e nei suoi dati strutturali più profondi. Forse è qui il nodo che ci trasciniamo, che combiniamo variamente nelle diverse finanziarie ed è un nodo che deve insieme camminare con un'ipotesi di sviluppo non crescente a livello europeo per il 2008 e con valutazioni del sistema complessivo, del sistema Paese di una non crescente produttività di sistema. Forse, se noi volessimo - al di là delle polemiche - assumere le riflessioni del ministro Padoa-Schioppa per quello che hanno voluto essere oggi pomeriggio,

forse, se volessimo tematizzare queste riflessioni e vedere da che parte aggredire il problema storico della improduttività di una spesa pubblica che è agli stessi livelli, se non superiori, per comparti, degli altri Paesi europei, metteremmo su gambe più tranquille la nostra stessa discussione. Non ritorno sui dati proposti dal relatore Legnini e dallo stesso ministro Padoa-Schioppa sulla sostanziale invarianza delle spese nel passaggio tra Camera e Senato,

che sono state tanto qui evocate, e faccio poi soltanto due riflessioni. Questa manovra, completa anche del decreto sul *welfare*, ha un impatto redistributivo

Questa manovra affronta problemi fondamentali che sono stati meglio affrontati dalla Camera: si pensi al rifinanziamento di fondi per la prima infanzia, o anche ai bilanci di genere, o ai fondi per l'ambiente; ci sono stati, nel passaggio da Senato a Camera, anche aggiustamenti puntuali necessari; ma l'effetto redistributivo complessivo non è altissimo, bensì medio; va apprezzato per quello che è: ci sono elementi di forte giustizia sociale, forti interventi sui redditi bassi, ma complessivamente è medio.

che il Gruppo Per le Autonomie in parte rappresenta, che sono per loro natura cruciali. La nostra valutazione è che la riforma della disciplina dell'IRES e dell'IRAP, specie per le piccole e medie imprese, sia di fatto un contributo importantissimo per lo sviluppo del tessuto produttivo del Nord. La nostra valutazione è che la manovra sull'ICI agevoli sensibilmente agevoli sensibilmente redditi e possibilità di circolazione dei medesimi in importanti aree del Paese. A nostro parere, l'estensione di quella che due anni fa fu la procedura proposta per la Pedemontana lombarda, vale a dire la possibilità di forme di associazione, di gestione anche in prima persona delle grandi infrastrutture compartecipate dalle Regioni, agevoli in forma sostanziale lo sviluppo del trasporto in grandi e decisive

Sud. Se avessimo la pazienza - naturalmente non posso farlo io: lo ha già fatto il relatore Legnini in dieci minuti - di comporre insieme i fattori nuovi di sviluppo e la sfida di razionalizzazione di spesa della manovra, a fronte anche di una diminuzione della pressione fiscale, penso ne risulterebbe che questa fiducia è meritata: la maggioranza propone ciò che era in grado realisticamente di proporre. Avrebbe potuto far meglio, specialmente forse per quanto riguarda la manovra sulle pensioni e i 10 miliardi di euro che vanno, anche giustamente, a beneficio di classi di età e di un vasta platea di lavoratori, ma vengono ovviamente tolti ad altri possibili interventi. Nella sostanza, però, nell'intimo, si tratta di una manovra che da una necessità politica ed economica ha affrontato quelle leve che non eravamo riusciti ad agire l'anno scorso e che in un quadro di tendenziale risanamento attuano anche elementi di sviluppo

Oltre certamente al cortesissimo sottosegretario Sartor, al relatore e a codesta Presidenza. Veramente ho una notevole difficoltà a trattare un tema che abbiamo già più volte visitato in Commissione e in Aula negli ultimi mesi, che è questo della trattazione della trattazione della stesura da parte del Parlamento di tutte le leggi indirizzate alla costruzione della politica economica e dei documenti finanziari per l'anno che viene; è una discussione che ci ha visti coinvolti tante volte, spesso su argomenti quanto più distinti possibile.

Fondo "per il potenziamento della ricerca e lo studio delle interazioni tra i fattori ambientali e la salute, sugli effetti che gli agenti inquinanti hanno sugli organismi viventi, e in special modo sull'uomo", eccetera, con una Fondo "per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio"; Fondo "per la promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, e climalteranti, nonché per la promozione della produzione di energia elettrica da solare termodinamico". Presidente, ma questi sono fondi che hanno un nome e un cognome,

vincolato dal proprio assetto ideologico, produce la finanziaria, dall'altro queste finanziarie che tutto sono tranne ciò che cercherò di dire nella chiosa finale politica al mio intervento.

ricavare allo Stato le risorse per bilanciare l'abbassamento del reddito sulle società qual è stato? L'impossibilità di considerare le spese per interessi superiori a una certa percentuale come oneri deducibili, cioè come oneri che possono essere imputati nella colonna dei costi dell'azienda. Ho cercato di spiegare che questo non avviene in nessuna parte del mondo anche perché l'investimento e, quindi, il trasporto - lo ho detto in Commissione più volte - dalla rendita al rischio del capitale non può essere un'opposizione, ma un'opportunità; e l'opportunità è data dal mercato, non può essere indirizzata dallo Stato. Ho cercato di dire che tutto questo aveva una giusta filosofia quando i tassi erano ben superiori al 6-7 per cento, che è il limite del rendimento dell'investimento proprio nelle aziende per alto valore aggiunto e, quindi, con una buona qualificazione produttiva.

bestiale. Mi sento di dover aggiungere che tutto questo viene coniugato con una filosofia che vorrebbe

l'equilibrio con la redistribuzione degli utili. Abbiamo già detto nel passato che una finanziaria - e, quindi, la politica economica - ha due obiettivi: la riallocazione delle risorse per favorire la produzione e la redistribuzione degli utili. Il problema sta nel ricercare l'equilibrio tra queste due manovre.

non preoccuparsi. Venendo al merito, sulla scorta delle valutazioni già ampiamente motivate nel corso della discussione svoltasi in prima lettura qui in Senato sulla legge finanziaria e sui provvedimenti ad essa collegati, non posso che ribadire l'apprezzamento per l'impianto equilibrato ed incisivo di misure le quali, pure in una condizione di forti condizionamenti e criticità, riescono efficacemente a contemperare rigore finanziario, sostegno allo sviluppo ed equità sociale. Un insieme di provvedimenti che, in coerenza con gli obbiettivi del programma presentato agli elettori, raccoglie i primi frutti dello sforzo di risanamento dei conti e si propone come supporto e stimolo al processo di ripresa dell'economia italiana che in questi 18 mesi ha già centrato importanti obbiettivi. I conti sono più in ordine, il *deficit* si riduce, il debito pubblico comincia a scendere

circa l'inadeguatezza di questa manovra di bilancio e anche molte dotte lezioni, con qualche citazione letteraria, su ciò che andava fatto per contenere di più la spesa, incidere maggiormente sul debito, ridurre la pressione fiscale. È un fuoco di sbarramento che con troppo disinvoltura evita di misurarsi con una doverosa assunzione di responsabilità a proposito di come la precedente maggioranza di Governo, tra cui tanti censori che abbiamo sentito oggi, ha consegnato l'Italia a questa XV legislatura. Ma è anche forse un modo di sfuggire al fatto di dover riconoscere che quello in esame è un buon disegno di legge e che in concreto questa manovra finanziaria dà corpo a risultati positivi difficilmente contestabili. Vorrei provare ad evidenziarlo assumendo l'ottica delle scelte operate sul terreno della politica fiscale, anche per trarne qualche valutazione sul lavoro compiuto e sul contributo, penso lo si possa dire, apportato dalla Commissione finanze e tesoro del Senato nel merito dei provvedimenti e dei contenuti. Penso in primo luogo alla questione della lotta all'evasione evasione e all'elusione fiscale: si tratta, come sappiamo, di uno dei capisaldi della politica economica e tributaria del Governo. Erodere con costanza ed incisività l'enorme evasione fiscale che contraddistingue il nostro Paese è la condizione per recuperare le risorse necessarie a ridurre la pressione fiscale sia sulle famiglie che sulle imprese. In questa direzione, come noto, i primi risultati non sono mancati e il recupero significativo di un extragettito ha già permesso di assumere misure sociali di rilevante portata verso le pensioni più basse e gli incapienti. Ma lo spazio per ulteriori recuperi di gettito è ancora molto ampio, come dimostrano i dati di recente forniti dalla Guardia di finanza, che ha saputo recuperare dalla lotta all'evasione ben 23 miliardi di euro di maggior gettito,

ma essi sono indubbiamente un riflesso dell'impulso che è venuto dall'azione del Governo e dall'indirizzo legislativo. E poiché la stessa tensione e lo stesso buon riscontro di attività e di risultati si registrano anche per l'Agenzia delle entrate e per l'attività di Equitalia, se ne può forse dedurre che veniamo da una stagione in cui qualcuno - aggiungete voi il nome - teneva, per così dire, il freno a mano tirato e non consentiva alla macchina di sprigionare tutto il suo potenziale rispetto agli obiettivi di lotta e di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale.

senza le quali il raggiungimento di analoghi risultati per l'anno prossimo avrebbe potuto essere messo a repentaglio. È questa impostazione di indirizzo politico generale, ma anche di conseguente traduzione in scelte coerenti, operative ed organizzative, che dà credibilità anche ad alcuni degli impegni più qualificanti inseriti nel disegno di legge finanziaria. Penso in particolare alle disposizioni dell'articolo 1, comma 4, che riprende proprio un emendamento elaborato dalla Commissione finanze e tesoro e oggi ulteriormente arricchito quanto a strumentazione di fattibilità nella versione definita dalla Camera dei deputati, in cui si stabilisce che tutte le eventuali maggiori entrate - dunque, come sottolineava il relatore Legnini, non solo quelle provenienti dalla lotta all'evasione fiscale - che dovessero realizzarsi nel 2008, eccedenti rispetto a quelle finalizzate al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, devono essere destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, attraverso l'incremento della detrazione d'imposta per i redditi da lavoro dipendente, da corrispondere attingendo ad un fondo appositamente costituito a tal fine, a decorrere dal periodo d'imposta 2008. Penso non sfugga a nessuno la rilevanza di questa determinazione, posto che la questione del potere d'acquisto dei salari è oggi nel nostro Paese un tema assolutamente critico, una grande questione sociale nazionale che sollecita appunto risposte appropriate. Proprio per questo, esprimo l'auspicio che sull'attuazione delle misure di riduzione del carico fiscale sui redditi da lavoro dipendente e su quelli assimilati, segnatamente le pensioni, ci sia una azione di controllo e di monitoraggio tale da rendere la disposizione di cui parliamo effettivamente efficace per l'anno d'imposta 2008, prevedendo altresì, dove possibile e sempre nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, un anticipo della revisione delle aliquote già nei primi mesi del 2008. Anche sul terreno della fiscalità la finanziaria contiene numerose e rilevanti novità positive che le modifiche introdotte alla Camera hanno ulteriormente affinato, prevedendo meccanismi di maggiore gradualità nell'entrata a regime del nuovo sistema IRES in una direzione, in una direzione, peraltro, già suggerita anche nel parere formulato dalla nostra Commissione, proprio per tenere conto delle esigenze complessive, ed anche della realtà delle piccole e medie imprese, che sono la forza ed il perno del nostro sistema produttivo. L'assetto del fisco, che esce da questa finanziaria, è per le imprese fortemente connotato nel senso della semplificazione e dello snellimento delle procedure e muovere nella logica di un profilo dell'imposizione come ausilio alla competitività, al rafforzamento dimensionale e patrimoniale, alla crescita. Il nuovo scenario di tassazione delle imprese, che consegue alle disposizioni della finanziaria, sia per l'IRES con l'aliquota che scende dal 33 al 27,5 per cento sia per l'IRAP con la riduzione dal 4,25 cento, potrà ovviamente incorporare ulteriori correzioni in corso d'opera ed assumere progressivamente una strutturazione ancor più precisa che ne registri al meglio il grado di sintonia con i profili e le caratteristiche di fondo dell'economia italiana e della variegata ricchezza delle sue tipologie di impresa. Ma è indubbio che esso, anche per effetto della graduazione, ove introdotta per la fase di transizione, migliori il quadro fiscale vigente e che pure opportunamente rimane invariato in alcuni punti significativi. Così pure è di straordinaria portata esemplificativa la misura che introduce un regime fiscale sostitutivo sui contribuenti minimi e marginali e che, proprio per la sua natura innovativa, richiederà - questa è una raccomandazione, sottosegretario Sartor - una azione costante di monitoraggio dell'attuazione della norma, anche in relazione al carattere opzionale del regime che è stato introdotto e che quindi dovrà essere sottoposto ad una verifica e ad una valutazione di efficacia e di coerenza con gli obiettivi prefissati. Infine, voglio sottolineare la positività della soluzione data con le disposizioni concernenti la scelta dei contribuenti di destinare il 5 per mille dell'imposta dovuta, che interpretano il senso dell'ordine del giorno approvato dall'Aula in occasione della discussione della finanziaria in prima lettura, anche grazie al forte impegno espresso dal nostro Gruppo proprio su tale questione. Non si può non valutare con soddisfazione l'incremento della dotazione finanziaria così conseguita, che offre garanzie precise, almeno per l'oggi e per il medio termine. Tuttavia rimane aperta la questione di pervenire, come lo stesso Governo ha convenuto, ad una messa a regime della facoltà per il contribuente e per l'istituto in sé, ampliandone anche l'efficacia in termini di risorse finanziarie e migliorandone la gestione. In particolare, si dovrà pervenire ad una drastica semplificazione ed accelerazione delle procedure di erogazione dei contributi ai soggetti ed agli enti aventi diritto, prevedendo eventualmente che il compito possa essere affidato direttamente alla stessa Agenzia delle entrate. Ma resta comunque il fatto - voglio darne atto - che proprio grazie a ciò che è stato previsto con la finanziaria in esame la prospettiva di portare a regime compiutamente questo aspetto appare oggi molto più vicina ed effettivamente concretizzabile. Per economia di tempo, non mi soffermo sulle molte altre disposizioni fiscali che realizzano effetti positivi sui bilanci delle famiglie e agiscono in difesa del loro potere di acquisto; penso alle detrazioni ICI sulla prima casa, all'ulteriore detrazione per le famiglie numerose, al corrispondente beneficio per chi non è proprietario e quindi se ne può giovare in termini di sgravio fiscale rispetto all'affitto, alla minore aliquota per il TFR, all'innalzamento del limite di detraibilità degli oneri per interessi passivi sui mutui per la prima casa, alla previsione di un meccanismo di sorveglianza dei prezzi degli alimenti ed alle norme a favore dei cittadini consumatori, che ora potranno far valere insieme le loro ragioni e chiedere il risarcimento in caso di lesione di diritti collettivi. Certo, signor Presidente, permangono difficoltà generali nel quadro socio-economico di prospettiva, così come tante ancora sono le questioni irrisolte o da migliorare e vecchi e nuovi problemi costituiscono ancora ostacoli ardui da superare. Tuttavia, questa finanziaria muove nella direzione giusta: riesce complessivamente a coniugare il risanamento e lo sviluppo con la giustizia sociale e indica la prospettiva di uno sviluppo, che si propone di essere inclusivo e che non vuole lasciare ai margini del diritto di cittadinanza le forze più deboli, i ceti più esposti alle criticità presenti nella nostra società. Per questo insieme di motivazioni sosteniamo convintamente la proposta di legge finanziaria e voteremo la fiducia al Governo, affinché questo possa agire per darvi attuazione nell'interesse del Paese.

La seduta è tolta